agli strumenti e modalità attraverso i quali avremmo poi dovuto attuare operativamente tutto il Piano. Questa carenza strategica è ancora più grave se consideriamo che una cifra importante, pari a ben 127 miliardi di euro sarà riconducibile a misure di indebitamento, che andranno a gravare sulle spalle del nostro Paese. Tutto ciò si traduce nell'affermazione di due concetti, uno conseguente all'altro: la totale assenza di progettualità e, conseguentemente,

delle misure che vengono rifinanziate tutti gli anni. Quest'anno è stata finanziata maggiormente, ma ci troviamo di fronte a una misura oserei dire

praticamente nulla. Si tratta di una materia sottostimata e sottoattenzionata, che non ha ricevuto risposte. C'è uno stato di asfissia, che sta paralizzando tutto il comparto, nei confronti del quale non arriva alcuna risposta, né tantomeno è arrivata in questa circostanza. Si è parlato dello sport in tutte le salse, ma abbiamo visto che, alla mancanza di un apposito Ministero, è stata contrapposta la presenza di un Sottosegretario, che non ha ancora presentato le linee operative

del mondo dello sport anche e soprattutto nel campo del dell'impiantistica sportiva. È stata data una risposta, che ritengo parziale, per quello che riguarda l'impiantistica sportiva, ma, rimanendo all'interno di questo campo, si poteva pensare di destinare risorse per l'abbattimento l'abbattimento dei canoni, o meglio per lo spostamento del pagamento dei canoni dell'impiantistica sportiva pubblica: stiamo parlando del 30 per cento degli impianti pubblici. Si poteva intervenire sul blocco dei distacchi

Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, ci stiamo occupando del Piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè del programma di investimenti che presenteremo all'Unione europea, per dettagliare il modo in cui pensiamo di spendere

Le risorse destinate all'Italia ammontano, come è noto, a più di 200 miliardi, di cui più di 80 a fondo perduto e oltre 120 sotto forma di prestiti. Ci troviamo, quindi, in una condizione forse irripetibile della storia del nostro Paese perché abbiamo finalmente le risorse finanziare e, sperabilmente, la volontà politica per costruire un'Italia nuova, cogliendo tutte le opportunità che derivano dalla transizione ecologica e digitale. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza si fonda e si snoda su tre assi strategici (la digitalizzazione e l'innovazione, la transizione ecologica e l'inclusione sociale) e tre priorità trasversali (la parità di genere, i giovani, il Sud e il riequilibrio territoriale). Tutto ciò corrisponde perfettamente ai capisaldi programmatici del MoVimento 5 Stelle sin dalla sua nascita. L'Italia deve diventare una protagonista assoluta del *green new deal* europeo e deve vincere la sfida della sostenibilità e della riduzione delle emissioni nei trasporti, nella produzione di beni e servizi, nella realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali. Ne siamo talmente convinti che per conseguire questo obiettivo abbiamo immaginato di creare un nuovo Dicastero (il Ministero della transizione ecologica), che accorpasse competenze che erano distribuite tra vari Ministeri e lo abbiamo posto come condizione per la nostra partecipazione al Governo Draghi. La sfida davanti a noi è grande e stimolante perché vogliamo costruire un'Italia diversa, nuova - come dicevo prima - più giusta, più inclusiva, più *smart*, più pronta al cambiamento, più rispettosa dell'ambiente e delle future generazioni. Perché tutto ciò accada occorre che il Piano nazionale sia accompagnato da una serie di riforme che il Paese aspetta da decenni - penso a quella dell'intero sistema tributario, del mercato del lavoro e alla riforma per velocizzare e rendere efficiente la macchina della giustizia e, infine, da tutte le misure volte a promuovere la concorrenza. Per l'Italia nuova che abbiamo in mente, per creare lavoro e benessere, per redistribuire ricchezza, abbiamo innanzitutto necessità di una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini digitalizzata, sburocratizzata, ben organizzata ed efficiente che non costituisca un fattore di ritardo negli investimenti pubblici e privati. Abbiamo bisogno che cittadini e imprese possano operare in un contesto di legalità che favorisca il merito e l'innovazione, che promuova lo sviluppo delle idee e della ricerca, che consenta di utilizzare al meglio le tecnologie. Tutto ciò deve aumentare la ricchezza del Paese e la produttività delle imprese, ma soprattutto deve migliorare la qualità della vita delle persone, che è e deve rimanere il nostro obiettivo prioritario. La transizione ecologica non deve essere uno *slogan* o il nome di un Ministero; non permetteremo di fare operazioni di *greenwashing* o di ecologismo di facciata, ma impegneremo tutte le nostre forze affinché la transizione ecologica e digitale, l'attenzione al Sud e il riequilibrio territoriale costituiscano uno straordinario e potente motore di nuovo sviluppo per far partire nuove filiere produttive, aumentare sensibilmente l'efficienza energetica del nostro complesso economico e aumentare la produzione di energia rinnovabile, ridurre drasticamente le emissioni di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria, dei nostri mari e dei corpi idrici. Per quanto riguarda l'inclusione sociale, territoriale e di genere, occorre intervenire sulle diseguaglianze e contrastare le diverse povertà, a partire da quella economica - abbiamo iniziato a farlo fin da subito con il reddito di cittadinanza, che questo Governo continua a finanziare, a riprova della bontà della misura, checché ne dicano gli amici degli evasori fiscali - e da quella culturale, migliorando l'istruzione e la trasmissione delle conoscenze, anche digitali, investendo massicciamente nella scuola pubblica. In merito alla parità di genere, è davvero tempo di porre in essere i provvedimenti che consentano di rimuovere tutti gli ostacoli che rendono alle donne difficili se non impossibili la formazione, il lavoro e l'accesso alle risorse finanziarie, che costituiscono nel loro complesso una vera e propria discriminazione che troppo spesso relega le donne al lavoro domestico e di cura privando l'Italia di talenti che, invece, hanno tutto il diritto di esprimersi e da cui il Paese trarrebbe enormi benefici. Se oggi possiamo parlare di tutto ciò, se possiamo parlare di 209 miliardi da investire, lo dobbiamo all'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte *(Applausi)* che, insieme al MoVimento 5 Stelle che lo ha sempre sostenuto,

Conte ha saputo cambiare l'Europa in pochi mesi, trasformando un insieme di Stati egoisti e fautori dell'*austerity* in una Unione pronta a fare cassa comune, a fare debito comune, ad aiutare finanziariamente chi ha più bisogno. Questa trasformazione è avvenuta a dispetto sia di alcuni soloni dell'informazione militante italiana sia di una opposizione becera, capace solo di dispensare insulti a piene mani e di sbagliare ogni previsione al riguardo. Oggi fa sorridere ripensare alle dichiarazioni roboanti e di bassa propaganda di qualche settimana fa di chi - come la Lega, ieri all'opposizione, oggi al Governo - sosteneva che l'Italia non avrebbe dovuto prendere nemmeno gli 80 miliardi che l'Europa aveva deciso (per noi, non certo per loro) di regalarci per superare la crisi economica, perché a loro dire non conveniva. Ora, invece, vogliono insegnarci come si spendono i 209 miliardi. Benvenuti nel mondo reale!

Piano nazionale di ripresa e resilienza: non si era mai visto nella storia della Repubblica italiana - dal Dopoguerra a oggi - un provvedimento così importante per la vita presente e futura della Nazione. Un documento programmatico di incredibile ampiezza, che vale quasi tre volte quel piano Marshall che fu messo in atto per risollevare il Paese dopo un conflitto mondiale: 209 miliardi. Insufficiente e deludente nella sua prima stesura, ora, con le osservazioni proposte dal Parlamento e con la revisione fatta da questo Governo, comincia a diventare un piano strutturato. Ci fanno molto piacere le dichiarazioni di ulteriore condivisione del Ministro dell'economia, che abbiamo letto sui giornali, perché abbiamo un'opportunità unica per rivoluzionare in senso virtuoso l'intero sistema Paese. Per questo servono visione, concretezza, coraggio, competenza, forza decisionale condivisa. Piano nazionale di ripresa e resilienza: vi prego di concentrarvi sui termini con cui è stato definito un piano che questo Governo e il Parlamento, che è la voce dei cittadini, hanno la responsabilità di realizzare. Per lavorare meglio dobbiamo concentrarci su ogni singola persona che, in quanto tale, ha diritto a realizzare la propria vita in serenità. E allora, E allora, mentre pensavo a come intervenire su questo Piano, ho visto e ho negli occhi l'impegno di un sanitario che lotta ogni giorno per salvare vite; vedo il sorriso di una cassiera alla propria postazione, sempre, dall'inizio; la pazienza di un genitore che si divide tra *smart working* e didattica a distanza; il calore dei volontari che confortano, che aiutano. Vedo la disperazione e la forza di un commerciante, di un imprenditore, di un agricoltore che cercano di resistere in ogni modo e si fidano e si affidano a noi. Ascolto gli sfoghi dei ragazzi a cui la pandemia ha tolto la vita sociale; sento gli sforzi decuplicati di chi assiste le persone anziane malate, disabili, all'interno della famiglia. E potrei andare avanti. Vedo quei bambini per cui l'unico pasto nutriente era quello della mensa scolastica, e sono sicura che voi li vedete con me e per questo siamo tutti protesi a fare il meglio possibile, spinti e ammirati da quella silenziosa, ma fortissima, dignità che ha caratterizzato il popolo italiano nel suo momento più duro. Ogni singola persona merita tutto il nostro sforzo per realizzare un Piano fatto bene, che è la più grande sfida che il Paese deve affrontare e vincere e dobbiamo farlo con amore. Bisogna fare bene e far tornare la fiducia; bisogna fare cose egregie, non solo per avere la sufficienza in Europa, ma per raggiungere l'eccellenza che questo Paese si merita. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza può farci entrare nella storia, dobbiamo scegliere se farlo da eroi o da perdenti. Noi vorremmo essere ricordati per essere riusciti a cambiare le cose; oggi gli italiani resisteranno e stringeranno i denti ancora un poco, se sapremo dare loro la certezza che i loro sacrifici saranno ripagati, se lasceremo lavorare chi vuole lavorare, se sapremo creare per tutti le condizioni di una vera ripartenza e queste condizioni si basano su due pilastri non negoziabili: fiducia e libertà; fiducia e libertà che devono stare alla base della grande alleanza tra pubblico e privato. Occorrono regole certe e semplici nella loro applicazione e di pari passo riforme, riforme e riforme. Serve un'opera rivoluzionaria, perché oggi questo Governo potrà decidere del futuro dell'Italia. Forza Italia c'è dal primo momento, impegnata al massimo per dare un contributo competente ed efficace secondo i principi liberali, riformisti, solidaristici e popolari che caratterizzano il nostro movimento. La transizione ecologica diventa centrale in questo lavoro e per Forza Italia lo sviluppo sostenibile non può prescindere dal sostegno all'innovazione tecnologica, nella convinzione che l'iniziativa privata sia da accompagnare, a partire dalla rigenerazione urbana, tema centrale per la ripartenza, perché la bellezza salverà il mondo,

libertà di scelta educativa, accompagnamento al rientro degli studenti che assicuri un sostegno agli insegnanti e ai docenti, revisione dei programmi per adeguarli al mondo che cambia. Siamo nati per ricominciare. Così mi ha detto ieri un collega, incidentalmente il Presidente della 6a Commissione. Vediamo di ricominciare alla grande, per un nuovo miracolo italiano.

che ridisegni davvero la geografia sociale di questo straordinario Paese e che venga utilizzato dall'Unione europea. Si tratta, infatti, di un Piano per l'Italia, per la Francia e per la Germania, ma costruito costruito dall'Unione europea per raggiungere un obiettivo che oggi si intravede, ma che non è certo possa essere raggiunto. La terza considerazione da fare è che implica un impegno

A differenza del passato, quando le pandemie come la peste erano considerate grandi livellatrici sociali, questa pandemia ha generato ulteriori diseguaglianze diseguaglianze che sono ruzzolate assieme a rancore e spesso al rancore non è seguita la speranza, come per i nostri nonni e i nostri padri all'indomani della seconda guerra mondiale, ma la rassegnazione. Pertanto il PNRR, su cui le Commissioni riunite 5a e 14a hanno fatto un ottimo lavoro, può sortire questi effetti alla sola condizione che crei uno Stato più umanitario e, dall'altra parte, metta l'Unione europea nella condizione di reggere la sfida competitiva tra Stati Uniti e Cina. C'è un *affidavit*, che noi abbiamo messo nelle mani del Governo più ampio che la storia della Repubblica abbia mai conosciuto e di un Presidente autorevole e decisamente europeista, non dell'ultima ora. Quando parlo di uno Stato più umanitario e, quindi, più inclusivo, che si impegni soprattutto a consentire garanzie e prospettive certe per le giovani generazioni e che metta l'Europa nella condizione di giocare una partita che, negli ultimi venti anni, ha cessato di giocare in maniera competitiva nel palcoscenico internazionale, parlo di una questione strategica, per la quale questo Paese e l'Europa esigono governanti strabici. Il PNRR non si governa con il presentismo, con la moda di questo tempo. C'è bisogno di profondità, c'è bisogno di strategia e c'è bisogno decisamente di lungimiranza. La seconda questione che sottolineo riguarda la centralità che è stata affidata al Parlamento. Ne prendo atto, è un fattore assolutamente positivo. Nel parere che le Commissioni hanno espresso, è sottolineata la questione riguardante non soltanto la giornata di oggi, ma soprattutto la fase successiva, con il coinvolgimento del Parlamento, da parte dell'Esecutivo, nella fase di concretizzazione delle proposte che verranno.

svuotare i cassetti, infilandoci progetti di qualsiasi natura, serve a metà e non modifica, né rovescia la storia. Ho letto attentamente soprattutto il piano delle infrastrutture, non soltanto quello che riguarda la Commissione che ho il privilegio di presiedere. Capisco il punto chiave sia consentire un forte sviluppo, l'accorciamento della differenza tra Nord e Sud - è evidente - e un forte sviluppo legato soprattutto alla piattaforma orizzontale del Nord Italia, che è la prima che si collega con forza, con tenacia e con determinazione al resto dell'Europa. Registro, però, all'interno del *recovery plan*, leggendo le proposte, anche una sorta di cesura fra il Nord e il Sud dell'Italia. L'Italia centrale non c'è

tra due pezzi del Paese. L'ultima questione riguarda il lavoro svolto dalla mia Commissione, del quale vado orgoglioso. Vi abbiamo inserito punti significativi, che riguardano il tema delle radici e delle identità dell'Italia di mezzo, investimenti sul merito, le tutele di persone più che di entità dimenticate. Abbiamo cercato di ricostruire di ricostruire un pilastro decisivo, che peraltro era già stato previsto e che noi abbiamo soltanto allargato, attorno a istruzione e ricerca. Istruzione e ricerca, accanto alla giustizia e alla salute, rappresentano uno dei tre pilastri attorno ai quali si costruiscono le Nazioni. In questo caso, l'ordinamento statale è stato chiaro: questi tre pilastri vanno protetti e salvaguardati e quello che noi abbiamo fatto è accrescerne le potenzialità.

all'evasione fiscale, con la gestualità del corpo, magari distrattamente (perché non voglio dire che l'abbiano fatto apposta: ci mancherebbe), indicano una parte dell'emiciclo, facendo intendere, a chi guarda in quel momento,

investimenti e riforme. È evidente che se vogliamo far ripartire il Paese, per esempio attraverso la parte infrastrutturale, non è possibile non pensare a una riforma del codice degli appalti, altrimenti ricominciamo ad essere quelli che dicono che ci sono 150 miliardi fermi e non riusciamo a utilizzarli. Voglio sottolineare il grande lavoro svolto dalla mia Commissione, un lavoro proficuo ha portato a trasmettere un parere alle Commissioni di competenza di 79 punti. Mi piace ricordarne alcuni: il consolidamento delle filiere decisive per l'industria nazionale, per esempio quella manifatturiera, attraverso la digitalizzazione. La nostra industria manifatturiera è *leader* a livello internazionale ed è sicuramente quella che in questa fase ha subìto più danni. Il nostro Paese è sicuramente succube e ha un *gap* fortissimo di dipendenza sulle materie prime: è evidente che va ridotto. Siamo in procinto di esaminare un affare assegnato, assieme alla 9a Commissione, proprio per parlare di questo: l'aumento dei prezzi. Forse si è deciso anche di convocare in audizione il Presidente cinese, ma vedremo. Vi è poi la richiesta fortissima di semplificazione dell'*iter* burocratico per l'ottenimento e l'installazione degli impianti fotovoltaici, così come quelli per il mini idroelettrico.

ma va detto con grande forza (spero che sia una battaglia della Lega), anche la parte della difformità edilizia, perché la difformità edilizia all'interno della partita del superbonus è determinante. La nostra storia ci dice infatti che ci sono molto spesso difformità tra lo stato di progetto e lo stato di fatto, che non necessariamente sono condoni, ma sono piccole difformità: un metro, due metri, una finestra,

Abbiamo anche inserito il fondamentale ruolo di ENIT, anche in questo caso attraverso la parte digitale, per creare collegamenti e relazioni per il comparto del turismo che ha subito una violenza economica da questa pandemia.

progetti, insieme alle riforme, e serve che tutto parta. Signora Presidente, mi scuso per lo sfogo iniziale, ma era doveroso rispondere: non mi sento un evasore fiscale. Concludo dicendo che questo Piano, finalmente alleggerito dalle posizioni ideologiche, ambientaliste e dei microcosmi che forse venivano

Ma, anche avendo a disposizione tutto il denaro necessario e una burocrazia ridotta ai minimi termini, il problema essenziale è umano: quante persone occorrono per portare avanti in contemporanea tutto ciò che è previsto? Le esperienze italiane direbbero che promuovere contemporaneamente diversi progetti significa non portarne completamente a conclusione nessuno. Siamo, però, tutti consapevoli delle opportunità che arrivano adesso dall'Europa, che non devono essere sprecate. Sappiamo che non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, nemmeno in contabilità e finanza, e il lavoro di queste settimane, in ogni Commissione, è stato svolto e mirato all'ascolto. Le proposte arrivate da più fronti rappresentano una speranza. Il nostro Paese vuole crescere ma, per farlo, sappiamo che molto deve cambiare, a partire dal processo di sburocratizzazione. Due delle sei missioni contenute nel *recovery plan* sono quelle su cui voglio soffermarmi: equità sociale e di genere e salute. Con riferimento al primo punto, nel quadro degli interventi è necessario investire in primo luogo e con decisione in politiche di prevenzione che, in linea con quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul, attraverso interventi sul piano dell'educazione, consentano di affrontare la questione culturale dalla quale si origina la violenza contro le donne. prevenzione culturale non può prescindere dall'inserimento nei piani triennali dei diversi istituti scolastici di specifici programmi sulla violenza di genere e sull'educazione al rispetto. È altrettanto essenziale intervenire su una formazione adeguata del corpo docente: solo se adeguatamente formati gli insegnanti sono in grado di trasmettere modelli educativi fondati sul rispetto dei sessi. È necessario investire nella partecipazione delle donne al mondo del lavoro, valorizzandone il contributo, ma una promozione sulla parità di genere non può prescindere dall'implementazione di tutte quelle misure atte a favorire l'equilibrio della conciliazione dei tempi e a sostenere i nuclei familiari monoparentali, costituiti da tante donne. Con riferimento alla sanità, il nostro Gruppo ha cercato di portare all'attenzione diverse tematiche che enumererò: che enumererò: ammodernare il parco tecnologico e digitale ospedaliero; incentivare l'innovazione farmaceutica nell'ambito delle malattie rare, con l'abrogazione di *payback* per farmaci orfani innovativi; incrementare la capienza del fondo dei farmaci innovativi oncologici e non oncologici in vista dell'arrivo di numerose terapie avanzate ad alto costo; promuovere e rafforzare l'assistenza di prossimità; istituire il fascicolo sanitario elettronico, cominciando con un sistema semplificato. È dal 2017 che parliamo di fascicolo sanitario elettronico, che avrebbe dovuto essere pronto a dicembre e ancora tante Regioni non ce l'hanno. Occorre, poi, finanziare un piano cardiocerebrovascolare, che assicuri una gestione tempestiva e appropriata delle patologie; ridisegnare la rete dell'assistenza ospedaliera, potenziando la struttura organizzativa dei reparti, per snellire le liste di attesa e recuperare il periodo di emergenza, con particolare riferimento ai pazienti oncologici e cardiopatici cronici. Occorre intervenire sui reparti di area critica, dalle sale operatorie alle terapie intensive, creando posti letto veri e non soltanto sulla carta, come è stato fatto ad agosto, quando c'erano i posti letto ma non c'era il personale per rendere il posto in terapia intensiva agibile; potenziare l'assistenza domiciliare con una rete territoriale integrata; rivedere la formazione del medico di famiglia e farne una specializzazione, come tutte le altre afferenti all'università; sostenere la fragilità, la cronicità, la disabilità; rivedere piani nazionali specifici obsoleti, non rinnovati nonostante lo preveda la legge che li ha istituiti; sostenere la fragilità ossea, vera emergenza di salute pubblica, superiore alla media europea; prevedere linee guida del Ministero per modelli multidisciplinari, come nel resto dell'Europa. Soprattutto serve un organo di vigilanza nel Ministero della salute, che controlli e vigili sui tavoli specifici, sollecitando il Ministro o chi per lui.

L'assistenza alla salute mentale: esiste uno scollamento tra i bisogni del paziente e le risposte del Sistema sanitario nazionale. I LEA devono essere aggiornati e aspettiamo ancora di Sono in aumento le forme depressive e i disturbi del comportamento alimentare: più di 3 milioni di ragazzi e ragazze muoiono per anoressia e non sanno a chi e dove rivolgersi. potenziare l'assistenza materna e infantile, perché potenziare le politiche demografiche significa ricondurle il più possibile al rispetto dei tempi di fecondità naturale di ogni donna. È stato un inizio un po' tortuoso, ma la partita è ancora da giocare. E spero che ogni processo possa essere trasparente nel modo reale della trasparenza - non inteso come tanti dicono,

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, Ministri, colleghe e colleghi, il nostro Paese sta attraversando un periodo difficile. L'Italia, come l'Europa e il mondo intero, è stata travolta da uno *tsunami* sanitario, che ha trascinato con sé la tenuta economica e sociale del nostro vivere civile. È doveroso quindi intervenire per porre rimedio a questa catastrofe e consentire la ripartenza del nostro Paese, come dell'Europa. Tuttavia, il Piano nazionale di ripresa e resilienza può costituire un'occasione storica per affrontare non solo l'emergenza sanitaria, ma anche, con decisione e interventi incisivi, altre crisi ben più gravi e antiche che attanagliano il nostro Paese. Una è la crisi ambientale, che riguarda il pianeta intero; l'altra è la disuguaglianza socio-economica tra i territori ed è specifica dell'Italia, che vive da troppo tempo il divario Nord-Sud.

Partiamo dagli interventi che riguardano più specificamente la transizione ecologica. In armonia con il parere espresso anche dalla Commissione di cui faccio parte, ritengo che all'agricoltura vada dato un maggior spazio, perché nessuna rivoluzione in senso ecologico può essere fatta senza dare il giusto risalto

assegnati esclusivamente a contratti di filiera, logistica e parchi, che però non incidono in modo significativo sulla transizione ecologica. Non si interviene - per esempio - sul ruolo svolto dalle aziende agricole, in particolare quelle zootecniche, nella prevalenza di modelli di produzione intensivi e dipendenti dall'uso di sostanze chimiche di sintesi, che hanno un elevato impatto sulle varie matrici ambientali. Su questi elementi occorre prevedere una strategia di intervento ben chiara, poiché oggi l'agricoltura intensiva sembrerebbe essere una delle cause di perdita della biodiversità in Italia e in Europa. In generale, l'unica agricoltura veramente amica di un nuovo modello di sviluppo verde è quella biologica, che ha peraltro un importante ruolo di potenziamento della prevenzione sanitaria e, quindi, consentirebbe anche di gravare meno sui sistemi sanitari nazionali. Inoltre, nel programma Next generation EU viene destinato il 37 per cento delle risorse alle azioni per il clima, all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla biodiversità terrestre e marina. Nel nostro PNRR, invece, il tema della tutela della biodiversità non viene affrontato concretamente con linee di intervento *ad hoc*. Sarebbe dunque necessario aggiungere al PNRR un capitolo su "Conservazione della biodiversità e restauro degli ecosistemi". Inoltre, la distribuzione delle risorse nell'ambito degli obiettivi appare discordante. mentre alla tutela del territorio dal rischio idrogeologico vengono assegnati solo 3,7 miliardi, appena l'1,6 per cento, e all'economia circolare solo il 2 La verità è che, nonostante la buona volontà dimostrata con il *green deal* europeo e con lo stesso Next generation EU, non riusciamo ancora a intravedere l'urgenza della catastrofe generata dalle attività umane. E, se siamo disposti a parlare di guerra e di mobilitazione straordinaria nel caso di Covid, sembriamo ancora troppo lenti nell'intraprendere con decisione la strada di un nuovo modello di sviluppo. sanità (OMS) ci dice che, negli ultimi quaranta anni, con il cambiamento climatico ci sono state circa 150.000 vittime l'anno. Secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), 22 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le loro terre L'altro tema importante è l'appiattimento degli squilibri territoriali. L'Unione europea ha tenuto conto di tre criteri: popolazione, tasso di disoccupazione e reddito. Il PNRR è tenuto a procedere in modo trasversale, nelle sei missioni che lo compongono, con la locazione territoriale degli investimenti rispettando i tre criteri. L'obiettivo minimo del 34 per cento appare ampiamente insufficiente. Il rischio concreto è che Bruxelles ci bocci il piano proprio perché non abbiamo rispettato questo criterio di fondo, applicato così chiaramente dalle autorità europee. È importante quindi che rispettiamo la locazione territoriale degli investimenti, i *target* di spesa, i risultati attesi... La politica ha quindi il compito di creare e diffondere condizioni di benessere, accelerare e supportare i processi virtuosi, dare risposta all'emergenza e ai bisogni della popolazione, soprattutto delle prossime generazioni. Abbiamo oggi un'occasione storica di tradurre questo principio in realtà e non dobbiamo sprecarlo. Signor Presidente, onorevoli colleghi e Governo, dopo lo tsunami pandemico dobbiamo ripartire, ma dobbiamo anche diventare più temprati alle avversità. Ripresa e resilienza - le due parole magiche del Piano che oggi discutiamo - devono reggersi su salute, giovani, coesione sociale, ricerca scientifica, innovazione, digitalizzazione, infrastrutture, tutela dell'ambiente e transizione ecologica. Dobbiamo rimettere in moto il Paese partendo dalla tutela dell'ambiente e dalla prevenzione dei rischi naturali, promuovendo la cosiddetta economia della conoscenza. Utilizziamo le informazioni per generare valore, secondo l'etica della sostenibilità, attendendo al benessere sociale e ambientale. Non solo PIL: il progresso - quello vero - deve attuarsi rispettando l'ambiente, prevenendo i rischi naturali, utilizzando fonti energetiche rinnovabili, adottando processi produttivi e stili di vita compatibili con le capacità dell'ecosistema di assorbire gli effetti delle attività umane. È proprio in questa logica che ho inteso presentare numerose proposte al Piano. Affinché si possa intraprendere una lotta integrata al degrado fisico e antropico dell'ambiente, si devono mettere a frutto tutte le competenze scientifiche, tecniche e professionali del nostro Paese e ripensare i modelli di *governance* in tema di tutela ambientale e governo del territorio, a livello nazionale e locale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione. Si devono pensare nuovi modelli operativi sinergici che gestiscano al meglio le risorse a nostra disposizione. Bisogna creare una rete tra le istituzioni sovranazionali, nazionali e territoriali, le agenzie governative, gli enti di ricerca e i privati perché si programmino gli interventi e non si gestiscano solo le emergenze. Ho così proposto che i Presidenti delle Regioni e i commissari straordinari contro il dissesto idrogeologico siano supportati da una struttura tecnica regionale dotata di uffici per lo studio, la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di difesa del suolo. molto importante prevenire i rischi ed è indubbio che il primo strumento di prevenzione sia la conoscenza. Si dia perciò spazio alla ricerca scientifica, geoscienze, energia, ambiente: è questo un grande progetto in tal senso; ricerca scientifica sul sistema terra, sulle fonti energetiche rinnovabili che il pianeta ci offre, sulle funzioni ecosistemiche dell'ambiente. Promozione delle attività conoscitive di prevenzione, nell'ottica di una corretta pianificazione territoriale e urbanistica, significa anche favorire il completamento e l'aggiornamento della cartografia geologica, dell'inventario dei fenomeni franosi italiani, ma soprattutto incrementare le scarse risorse annunciate per il contrasto al dissesto idrogeologico. Così come previsto, serve circa un secolo per completare la difesa del suolo; più realisticamente, saremo sempre a rincorrere le emergenze tra morti, distruzioni e lacrime di coccodrillo. Occorre investire non meno di 8 miliardi di euro in aggiunta a quelli in essere; il totale diventerà solo il 25 per cento dei 44 miliardi complessivamente necessari, ma ci permette di centrare pragmaticamente l'obiettivo della sicurezza idrogeologica in venticinque anni, intervenendo secondo le necessarie priorità. Gli investimenti in questo settore, oltre che strategici, saranno un moltiplicatore keynesiano, considerato che l'emergenza idrogeologica costa cinque volte di più della prevenzione. Al rischio idrogeologico occorre aggiungere l'elevato rischio sismico, il fabbisogno energetico, l'inquinamento ambientale. Ho quindi proposto di incrementare il fondo per l'adeguamento sismico degli edifici pubblici - in Italia abbiamo 13.200 scuole che non sono sicure e per incentivare l'edilizia residenziale, che si adegua ad una pericolosità maggiore a quella prevista dalle norme vigenti, in modo da salvaguardare, oltre che la vita, anche gli edifici. Vi ricordo che la ricostruzione *post* sisma vale l'85 per cento del costo di un terremoto: 36 miliardi di euro negli ultimi tre grandi terremoti in dodici anni. Qui il moltiplicatore keynesiano può diventare dieci necessaria la forestazione urbana di Città metropolitane, capoluoghi di Provincia o comunque di tutte le città più inquinate. È il caso di favorire, tra le fonti energetiche rinnovabili, quelle meno impattanti per l'ambiente e il paesaggio paesaggio - non trascuriamo la bellezza - fotovoltaico sui tetti, microeolico, geotermia a bassa entalpia, idroelettrico ad acqua fluente, idrogeno verde. Ho poi sostenuto la necessità di attivare progetti di*smart precision farming* per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie abilitanti dell'Industria 4.0, per la promozione del settore agricolo e per una sua sostenibilità ambientale. Infine, ho proposto che il Servizio sanitario nazionale garantisca i livelli minimi di assistenza per la cura e la prevenzione, innanzitutto, delle dipendenze patologiche. patologiche. Da oggi queste proposte sono linee guida per il Governo e auspico che si trasformino in azione per quel necessario futuro prospero, sereno e sostenibile che la Nazione merita. *Sursum corda*! Che la politica si doti di quel necessario coraggio che questo momento epocale richiede; un coraggio sostenuto dall'amore per il prossimo, per le future generazioni e per l'Italia.

mi preme partire da alcuni semplici principi di igiene del dibattito, che poi non sono altro che il riconoscere la grande varietà di sfumature che ha il nostro lessico. Se ci sono parole diverse, sarà per indicare concetti diversi: ad esempio, "maggioranza" non è "unanimità"; "unanimità" non deve necessariamente essere "conformismo"; "conformismo" forse è un po' più cugino di "piattume", che è abbastanza fratello di "squallore". Una cosa particolarmente apprezzabile nel discorso che il signor Presidente del Consiglio fece quando si presentò a queste Camere fu l'affermazione che nessuno dei partecipanti al progetto di questo Governo avrebbe dovuto rinunciare alla propria identità. Era un'affermazione particolarmente intelligente, perché lasciava presupporre che si sarebbero valorizzati i contributi, anche critici. Infatti, si può essere critici nel sostenere un progetto - lo si può perché si apporta un contributo di analisi - e poi naturalmente ci si conforma alle decisioni della maggioranza nel nome di un interesse superiore.

a constatare che esiste un atteggiamento un po' piagnone del Parlamento, che lamenta di essere conculcato dal Governo, ma poi, quando si tratta di far valere le proprie prerogative,

innanzitutto, da una frase che tutti credo apprezzammo, perché era di buon senso, nel discorso del signor Presidente del Consiglio. Cito testualmente, scusandomi se leggo, ma la mia memoria ormai è quella di un anziano: «La quota di prestiti aggiuntivi che richiederemo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

Avevo inteso, in questa frase, che a me sembrava abbastanza esplicita, del signor Presidente del Consiglio, che egli intendesse dire che, siccome i prestiti del *recovery fund* sono debiti del nostro Stato e il nostro è uno Stato abbastanza indebitato, ci sarebbe stata una valutazione quantomeno sulla convenienza. Qui fideisticamente si assume che indebitarsi con la Commissione sia necessariamente più conveniente che indebitarsi con i mercati. Può anche darsi che lo sia, almeno nella dimensione molto limitata del tasso di interesse, ma la convenienza di un prestito ha tante sfaccettature e, quindi, le parole del signor Presidente del Consiglio mi sembravano particolarmente sagge.

dall'acribia, dall'acrimonia, quasi dall'acredine con cui nelle Commissioni riunite, sia al Senato che alla Camera, si è eliminato qualsiasi possibile riferimento alla possibilità di valutare la convenienza dei prestiti erogati dal *recovery* rispetto alla convenienza dei prestiti disponibili sul mercato. La richiesta della Lega era semplicemente di fare una valutazione.

l'Italia finora è l'unico Paese che ha dichiarato di voler accedere a quei fondi. Questo, dal punto di vista del mercato, è il segnale che l'Italia pensa di avere bisogno di una forma di prestito particolarmente agevolato, cioè indirettamente pensa che sul mercato troverebbe delle condizioni peggiori. Questa - lo dico veramente con tutto il cuore e senza voler criticare nessuno - è una ammissione abbastanza pericolosa, perché rischia di generare

punto. Prima, dal lato dei puri, mi è giunta la parola "regalo", ci avrebbero regalato non so quanti miliardi. miliardi. Se è un regalo, desidero capire come mai la Corte costituzionale tedesca il 30 marzo ha detto «No, grazie». noi vogliamo bene non tanto perché ci ricorda che esiste il diritto, quanto perché ci fa divertire, è pittoresca con quelle meravigliose toghe rosse. Sono dieci anni che la letteratura scientifica ha appurato che non dobbiamo preoccuparci.

rivendicando la nostra primazia sulla Camera bassa, diciamo che la loro prima Camera è il Senato - ha aggiornato al 13 aprile la discussione sulla ratifica delle risorse proprie,

Ma, finché non le vuole la Germania, dobbiamo stare attenti alla strada che scegliamo - in termini sia di comunicazione che di sostanza - nell'impostare una partecipazione e una comunicazione su questo progetto. Dico questo perché - lo ricordo ancora una volta - quando noi siamo realisti, vinciamo anche come Stato nazionale. Torno a dire che - secondo me - il fatto che dal 24 marzo la *web tax* in Italia sia sostanzialmente operativa, perché finalmente normata da una circolare dell'Agenzia delle entrate un dato, questo, passato abbastanza sotto silenzio sui *media* - è una vittoria significativa dello Stato di diritto, della capacità di un Parlamento e di uno Stato, nella sua sovranità (parola che esiste nella Costituzione), di impostare un rapporto sano verso delle realtà economiche anche sovranazionali e di dimensioni ragguardevoli. Il problema è che perdiamo quando siamo più realisti del re, ossia quando andiamo spesso a ratificare in anticipo e corriamo sempre avanti agli stimoli che ci vengono

Signor Presidente, mi consenta anzitutto di ringraziare i relatori per lo sforzo che hanno compiuto e ricordare che siamo in una discussione generale particolare.

di più lungo periodo e di inquadramento per avere esattamente la dimensione della sfida che abbiamo davanti. Vorrei soffermarmi solo su due snodi problematici e fare due raccomandazioni. Gli snodi problematici sono l'Europa e le riforme interne, forse i due pilastri di questo documento. Credo che l'Europa nel Secondo dopoguerra non sia stata

dopo il periodo bellico e a coinvolgere la forza economica della Germania nel momento nel quale la guerra fredda scalava uno dei suoi picchi più importanti. È stata l'Europa della CECA e poi del Mercato europeo In quel caso l'Italia fece la scelta giusta di fronte a quell'Europa pragmatica. Agganciarsi all'Europa, infatti, per un Paese che aveva subito poco prima la resa incondizionata, significò una cosa che fino ad allora la storia non aveva proposto a nessun popolo: popolo: rientrare nel consesso internazionale. Soprattutto, consentì all'economia italiana di depurarsi di quel velo di autarchia che le derivava dalla stagione precedente.

Fu una vera e propria rivoluzione, portata avanti da un uomo che si chiamava Alcide De Gasperi e da una formula politica che si chiamava centrismo. Un'Italia che era arretrata e fondamentalmente agricola, nel giro di pochi anni diventò una potenza europea e una potenza industriale. È questo il periodo che va

una pubblicazione di cui leggo una citazione: «Senza pretesa di esaustività, elenco le riforme più evidenti: rafforzamento competitivo dell'industria privata e pubblica; miglioramento della qualità della pubblica amministrazione in generale, di giustizia, scuola, università e ricerca in particolare; completamento e continuo aggiornamento di un programma razionale di infrastrutturazione e logistica; una politica efficace, coerente continua nei confronti della questione meridionale; un disegno di riduzione della dipendenza energetica; la fondazione di un sistema di *welfare* equo e sostenibile nel lungo periodo». periodo». Sembrano le riforme che abbiamo di fronte. Questa è un'analisi di Michele Salvati, un economista di sinistra, che fa l'elenco delle riforme mancate durante la stagione che viene chiamata del lungo centro-sinistra, che inizia nella metà degli anni Sessanta e finisce nella metà degli anni Novanta. Se ci aggiungiamo un po' di digitalizzazione e un po' di transizione ecologica, è il programma che abbiamo davanti.

condizionato stagioni successive, come quelle che vanno sotto il nome di seconda Repubblica. Hanno portato a un debito pubblico sproporzionato, a una fiscalità oppressiva, a un aumento delle divisioni

più, tra aree interne e coste. Abbiamo infatti, sulla dorsale appenninica, un Paese che si sta spopolando, in cui restano solamente alcuni dei borghi più belli d'Europa, dove c'è un'anima della nostra tradizione, assolutamente abbandonati. Di questi macigni e di queste riforme non fatte non ci siamo mai liberati. La fase che va sotto il nome di globalizzazione ha accentuato il peso di tutto ciò, ha comportato che il nostro Paese abbia una crescita più lenta - è un dato di fatto - di tutti gli altri Paesi europei dello stesso rango e poi ha provocato l'espulsione dal mercato di una parte della nostra impresa, che non è riuscita a compiere il salto da piccola impresa a impresa media, in qualche modo vanificando quello che era accaduto negli anni Ottanta, con l'esplosione del cosiddetto esercito delle partite IVA. Signori rappresentanti del Governo, vorrei che avessimo la consapevolezza che questa crisi pandemica è una grande opportunità, perché è una crisi globale, che ci dà la possibilità di scrivere su una lavagna bianca, che dà all'Europa la possibilità di riformarsi tornando ad essere un'opportunità e non un'oppressione burocratica, che dà all'Europa la possibilità di revisionare il Trattato di Maastricht, sia sul versante del patto di stabilità, sia sul versante del fiscal compact. Questa crisi, proprio perché è globale, relativizza anche i *gap* storici dell'Italia che si sono consolidati nel lungo periodo. Signori del Governo, spero che abbiate la consapevolezza che, se non fosse stata una crisi globale, tutti gli scostamenti che abbiamo fatto finora sarebbero stati

Con molta sincerità, sul versante della pandemia, anche per contingenze sfavorevoli, questo cambio di passo non si vede. Noi, signori del Governo, ci aspettiamo che sul *recovery* ci sia invece un'assunzione di consapevolezza e responsabilità che porti

va al Parlamento, a noi, affinché controlli il Governo, questa ambizione, e non si limiti a rivendicare un ruolo corporativo di mera partecipazione o di copartecipazione alle risorse. Di consociativismo si può morire. Noi abbiamo bisogno di un Parlamento che sferzi il Governo e non che chieda una piccola parte in commedia. *(Applausi)*. PRESIDENTE. Signor Presidente, Ministri, colleghi, a fine aprile il nostro Paese sarà chiamato a compiere un primo fondamentale passo verso quella che sarà l'Italia del futuro. Con la presentazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza ci assumiamo la responsabilità enorme di affrontare una sfida storica, che, se ben giocata, potrà cambiare la vita degli italiani. Molteplici e complessi sono gli obiettivi da raggiungere e troppi per essere ripercorsi nei pochi minuti che ho a disposizione. Per tale motivo mi soffermerò su ciò che considero l'obiettivo primario del Piano: la riduzione del divario tra Nord e Sud Italia; un divario talmente grande e difficile da colmare che ha fatto sì che il nostro Paese fosse il primo destinatario in termini quantitativi delle risorse del Next generation EU. Ministro, dobbiamo avviare un progetto che possa garantire a tutti i cittadini italiani, da Pantelleria a Bolzano, pari pari condizioni di partenza e pari opportunità affinché l'eguaglianza sia non solo formale, ma anche sostanziale. È necessario avviare con determinazione un cammino che permetta a chi vive al Sud di poter godere dei medesimi servizi di chi risiede al Nord (trasporti, sanità, asili nido, scuole assistenza agli anziani), di poter trovare e mantenere con la stessa facilità un lavoro, di riuscire a investire e a creare occupazione più agevolmente. Siamo consapevoli che da solo il Piano non basta, ma la questione meridionale è nazionale pertanto, serve uno sforzo di lungo periodo che vada ben oltre il 2026, anno entro cui gli interventi previsti dal Piano nazionale dovranno essere completati. Serve una strategia complessiva di politica economica che richiederà riforme strutturali incisive e fiscalità di sviluppo mirata, oltre che ovviamente progettualità, efficienza e velocità nell'utilizzo dei fondi strutturali europei e, soprattutto, di quel Fondo di sviluppo e coesione a oggi scarsamente utilizzato e che, invece, dovrà essere indirizzato all'80 per cento verso le Regioni per cui è stato ideato. Ministro, per questi motivi ho chiesto e ottenuto che nella proposta di Piano a breve in votazione fosse chiaro che la rapida cantierabilità delle infrastrutture -condizione necessaria per accedere alle risorse del *recovery* *fund* - non impedisse la progettualità di ulteriori opere necessarie a rifondare un Mezzogiorno dei diritti dello sviluppo e del lavoro. Tra tutte queste opere penso al collegamento stabile sullo Stretto di Messina, collegamento che purtroppo con amarezza ho notato rimanere per alcune forze politiche un vero e proprio tabù.

per motivazioni meramente ideologiche riconducibili al nostro *leader* Silvio Berlusconi, che con determinazione ha lavorato per la realizzazione di quest'opera ritenendola, come tutti noi, un'enorme fonte di opportunità. *(Applausi)*. Un'infrastruttura strategica per il nostro Paese e per la riaffermazione della sua centralità nel Mediterraneo. A questo scopo, sempre nella proposta di Piano oggi in discussione, abbiamo chiesto di tenere conto almeno dello studio sull'argomento dell'apposita commissione di tecnici ed esperti, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal precedente Governo. Uno studio che attendiamo ci venga trasmesso al più presto dal ministro Giovannini, al quale rinnoviamo la richiesta di poterlo visionare, e che secondo i ben informati sarebbe a sostegno dell'importanza di realizzare un collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Non vorremmo infatti che la commissione in questione, Ministro, avesse lavorato a vuoto, che la sua istituzione fosse stata una semplice scusa, un semplice *escamotage* per prendere - o peggio perdere tempo e che il documento elaborato dopo quasi un anno di lavoro si rivelasse solo cartastraccia. Lo dico al Governo, ai miei colleghi: le grandi opere sono possibili anche al Sud; non dobbiamo cercare alibi, ma trovare il coraggio e la volontà di avviarle. Nell'attesa di poter, quindi, vedere questo *dossier*, ho chiesto che i fondi del *recovery fund*, oltre che per la realizzazione dell'alta velocità fino a Reggio e la modernizzazione e implementazione della rete ferroviaria in Sicilia, possano essere destinati anche al potenziamento ed efficientamento dell'attuale sistema di attraversamento dello Stretto. Certamente sarà fondamentale capire quali e quanti progetti il Piano destinerà alle Regioni meridionali. Il ministro Carfagna ci ha assicurato che sarà introdotto un capitolo espressamente dedicato al Sud e che somme ingenti saranno riservate alla realizzazione delle infrastrutture; ne siamo lieti. Per questo ho ritenuto necessario inserire tra le proposte di Forza Italia poi accolte nel documento oggi in esame - che per ogni missione, per ogni progetto di investimento, le risorse destinate al Sud siano chiaramente indicate e chiaramente verificabili. Nel complesso la quota da destinare al Mezzogiorno non dovrà essere minore del 34 per cento del totale delle risorse che arriveranno dall'Europa, non per ridurre la questione a una percentuale di bandiera - attenzione! - né tantomeno a una mera logica rivendicazionista, ma perché dietro ai numeri, dietro alle statistiche che raccontano un'arretratezza economica, resa ancora più grave dalla pandemia, c'è la sofferenza vera che la gente vive quotidianamente sulla propria pelle. Manca davvero poco, Ministro, alla definizione del Piano; mi auguro che il Governo faccia tesoro di queste mie proposte e lavori per un'autentica coesione sociale e territoriale per consegnare ai giovani, quella *next generation*, di cui stiamo parlando, un'Italia migliore e più giusta. rappresentanti del Governo, il PNRR è il cardine del progetto che, accanto agli strumenti di programmazione economica, consentirà la ripartenza del nostro Paese. Una ripartenza che può essere concreta solo se sapremo associare alle linee di azione progetti all'altezza del programma europeo, per valorizzare davvero il potenziale di crescita della nostra Italia, colmando il divario territoriale con un'inversione di rotta, però, che parte proprio dal Sud. Delle sei missioni mi soffermo brevemente sulla numero 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) che, almeno nella proposta, lega il sistema infrastrutturale agli obiettivi del *green deal* nell'ambito della manutenzione stradale 4.0 per conservare nel tempo le caratteristiche funzionali delle strade urbane ed extraurbane e che, grazie a sistemi innovativi, potrebbe rappresentare il motore di un processo produttivo per professionisti e piccole medie e imprese, soprattutto a livello locale, dell'intermodalità e logistica integrata, per restare competitivi sul mercato riducendo il costo generalizzato del trasporto, per sfruttare le opportunità derivanti dai servizi logistici, abbattendo i costi per gli operatori della logistica e aumentando i benefici per lo Stato, riducendo anche le emissioni di gas climalteranti. corretto poi pensare finalmente ad un'alta velocità ferroviaria, che sia però vera e uguale per tutto il Paese; per far questo però è fondamentale superare qualificazioni fuorvianti dell'Alta velocità, come l'accezione *light* o confonderla con la semplice velocizzazione, e pianificare invece azioni e progetti che consentano non solo una riduzione dei tempi di percorrenza, ma anche stessi servizi per tutte le tratte con vetture adeguate e di garantire viaggi confortevoli e sicuri. L'Alta velocità per il Mezzogiorno non può essere solo annunciata, deve essere contestualizzata sui territori. È fondamentale comprendere che la rete ferroviaria veloce è possibile solo se, superando ogni barriera, riusciamo a completare il corridoio scandinavo-mediterraneo, che costituisce una ramificazione necessaria per i collegamenti da

un'opera strategica che permetterebbe di rendere economicamente sostenibili gli investimenti necessari per le grandi infrastrutture, come appunto l'Alta velocità. Solo così si può pensare di valorizzare anche il ruolo dei porti italiani, di intercettare i traffici merci intercontinentali e per il Sud prevedere interventi specifici per l'intermodalità e la logistica integrata nei porti di Augusta, Gioia Tauro, Taranto e Napoli, per potenziare il ramo occidentale di quel corridoio scandinavo-mediterraneo per le merci, collegare alla rete centrale gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Trapani per lo sviluppo di attività crocieristiche e attrarre investimenti delle grandi compagnie aeree per muovere grandi flussi di persone da tutto il mondo. Vorrei fare un breve accenno anche alla missione 1 sulla digitalizzazione, considerato che il settore della mobilità è fortemente interessato dal fenomeno dello sviluppo di nuovi strumenti tecnologici, la cui implementazione ci consente di avere degli obiettivi misurabili in termini di aumento della competitività dei trasporti e della logistica, unitamente alla crescita economica, sviluppo e occupazione con investimenti per sviluppare le infrastrutture digitali, garantire l'accesso ad Internet su tutto il territorio nazionale, estendendolo in banda ultralarga, incentivando l'uso della fibra, di nuove tecnologie, di 5G e ponti radio per le aree non raggiungibili. Occorre soprattutto collaborare con l'Europa per incentivare l'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale e il *cloud*, abilitando l'innovazione, riducendo lo spreco di risorse e aumentando sostenibilità ambientale e sicurezza. Se con il PNRR si avvieranno progetti validi, lo *shock* economico favorito dal superamento del *gap* infrastrutturale tra i territori consentirà la crescita generale per sostenere il debito pubblico del passato e quello per cui ci impegniamo con il *recovery Dobbiamo raccogliere la sfida della competizione globale, dimostrando al mondo che con l'enorme patrimonio di civiltà, di valori e di eccellenze che possediamo si può superare il *deficit* e armonizzare lo sviluppo con la legalità, l'efficienza della pubblica amministrazione, l'uso ragionato delle risorse e la tutela dell'ambiente. È una sfida che, riprendendo le parole di San Francesco d'Assisi, cominciando a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, all'improvviso ci sorprenderà a fare l'impossibile. È iscritto a parlare il senatore Errani. Ne ha facoltà. il *recovery plan* al piano Marshall. In effetti in parte è così, almeno per quanto riguarda la cesura nella storia, l'apertura di un altro capitolo che con il piano Marshall si realizzò allora nel Dopoguerra italiano e che con questo *recovery plan* si sta realizzando oggi in Europa - e io dico nel mondo - spesso nella inconsapevolezza proprio dell'Italia. Allora il piano Marshall non fu soltanto un piano di ricostruzione economica, ma di ricostruzione nazionale, che delineò la forma dello Stato democratico di allora e le sue capacità d'intervento interno ed esterno. Fu la base dell'Alleanza atlantica; fu la base del Piano casa di Fanfani, delle autostrade, dell'industria dell'auto italiana come capofila dell'industria italiana. Allora vi era la consapevolezza di quello che stava accadendo e di come l'Italia poteva riprendere un ruolo nel mondo. Oggi manca l'adeguata visione. Non vi è la visione di quello che l'Italia sta affrontando e di come deve affrontarlo. Ieri è stato evidente a tutti che nel partito di maggioranza relativa di oggi non vi è quella visione e, quindi, non vi è nel Governo. E dove si nota? Si nota in quello che ha detto Grillo nel suo *blog* (o, meglio, ha fatto scrivere Grillo nel suo *blog*) rispetto a quello che ha detto Di Maio in Commissione esteri. È come se nella Democrazia Cristiana di allora vi fosse chi lodava Washington e chi si asserviva a Mosca. Questa contraddizione fa parte del *recovery plan* nella sua collocazione di ricostruzione europea e italiana. Manca quella visione di europeisti e di atlantisti perché orgogliosamente patrioti. Noi, che siamo una forza di destra, siamo infatti patrioti e, di conseguenza, in quanto patrioti italiani siamo europeisti atlantisti. Non si può essere adeguatamente europeisti ed atlantisti se non si è prima patrioti, perché sta nell'identità italiana la natura dell'Europa e dell'Atlantico, cioè dell'Occidente. Senza quella identità italiana, non ci sarebbe stata - e non c'è - l'Europa e nemmeno l'Occidente. Questa consapevolezza ci deve muovere per realizzare, attraverso il *recovery plan*, un nuovo progetto nazionale e un nuovo Stato, che non sia lo Stato interventista di allora, ma che sia uno Stato stratega, cioè, di delineare gli scenari che, di volta in volta, si possono realizzare attraverso gli strumenti pubblici, le norme, gli accordi internazionali, così come le risorse da investire. Come devono realizzarsi, oggi, uno Stato stratega e l'Italia del futuro?

e l'energia verde sono i campi in cui l'Italia può disegnare una nuova *leadership* nel Mediterraneo, in Europa e a livello globale. Ci vogliono, però, gli atti conseguenti: per esempio, la rete a banda larga a controllo pubblico; per esempio, gli accordi bilaterali per la connessione dei cavi marittimi; per esempio, il recupero della dorsale a banda larga europea che ci apparteneva. la visione è un'utopia che non si realizza ogni giorno. In conclusione, certamente si devono difendere le filiere industriali: ma quali? Laddove vi sono aziende italiane e, di conseguenza, filiere che possono diventare oggi campioni europei. La cantieristica, lo spazio, la siderurgia, l'auto. Non si può lasciare l'auto a un campione europeo in cui non vi sia una presenza dello Stato italiano al pari dello Stato francese. È così che si ridisegna la visione strategica di una Nazione, che recuperi i tre grandi divari, ricostruendo la comunità nazionale che oggi manca. Il divario che si è ampliato tra Nord e Sud; il divario tra ricchi e poveri; il divario tra giovani e anziani. Una comunità, oggi, più che mai è la Nazione. Nel mondo globale, la Nazione si disegna se è anche una comunità: altrimenti, non è più nulla! Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, un fattore positivo che vedo nel testo prodotto dalle Commissioni è quando, nella parte iniziale, si prova a includere lo sforzo economico e di investimenti del Next generation EU in un quadro più ampio di investimenti pubblici che nei prossimi anni bisognerà concretizzare. C'è il Next generation EU, c'è il Piano nazionale, ma ci sono i fondi di bilancio 2021-2026, c'è il React-EU, ci sono i Fondi di coesione. Preciso questo, perché dobbiamo spiegare bene a noi stessi e agli italiani che non tutto quel che si farà nei prossimi anni è Next generation EU e che, oltre quello, c'è tanto altro da fare per far riprendere l'economia. C'è un dato su cui insisto da sempre ed è la misurabilità matematica di quel che faremo. Saremo giudicati in Saremo giudicati in modo oggettivo, neutro e non soggettivo, da un parametro che sarà appunto misurabile e in quanto tale non smentibile. tornerò in conclusione. Il mio intervento verterà sul tema delle infrastrutture, in particolare sulla missione 3, nonostante vi siano infrastrutture importanti anche in altre missioni. Prendo ad esempio la missione 2, laddove si interverrà bene sulle infrastrutture idriche, sulle dighe, sui depuratori, sulle reti idriche e fognanti, sulla grande adduzione e anche, forse in modo insufficiente, sul dissesto idrogeologico. Su questo tema, come ho avuto modo di dire durante l'audizione del ministro Giovannini in Commissione, c'è un problema oggettivo di coordinamento di tre Ministeri che intervengono nella gestione risorsa idrica: il Mit, che oggi si chiama diversamente, il Ministero per la transizione ecologica e quello per le politiche agricole. È necessario uno sforzo importante di coordinamento. Il grosso delle infrastrutture è nella missione 3. Parliamo di oltre 30 miliardi di euro: 28,3 per l'Alta velocità ferroviaria, un altro per la manutenzione stradale, 3,68 miliardi di euro per l'intermodalità e la logistica integrata. si parla finalmente di Alta velocità nel Mezzogiorno con due opere importantissime: la Salerno-Reggio Calabria, che a me piace definire la "longitudinale", e la "trasversale" o "diagonale" Taranto-Potenza-Battipaglia. In questo modo si chiude una rete dell'Alta velocità nel Mezzogiorno che fa - devo dire - giustizia in termini di civiltà, di democrazia e di sostenibilità sociale. Il Sud doveva avere l'Alta velocità e finalmente ci si avvia per realizzarla. Poi - ma questa è una mia opinione personale e spero che la Commissione che insediammo nel Conte-II al Ministero dia questo risultato - penso che questo disegno vada completato con l'attraversamento veloce dello Stretto con il ponte, in modo tale che anche gli investimenti ferroviari che stiamo realizzando in Sicilia abbiano una continuità con ciò che accade nel resto dell'Italia. La scelta dell'Alta velocità, oltre che essere un fatto di giustizia, di sostenibilità e di inclusione, è anche una scelta completamente coerente col *green deal* europeo e fortemente coerente - questo lo voglio rivendicare - con il lavoro dei Governi della scorsa legislatura. La "cura del ferro" e il documento Connettere l'Italia

Importante la nomina dei commissari, in maniera particolare perché si è scelto il nome dell'amministratore delegato di RFI, quindi il vertice massimo della società pubblica che deve realizzare l'opera. Però, l'insistere sui commissari non deve far venir meno l'obiettivo principale, che è realizzare opere in questo Paese senza ricorrere a commissari, senza ricorrere a deroghe, senza ricorrere di volta in volta ad artifici. Bisogna rimettere mano - lo ministro Giovannini - alla reingegnerizzazione di tutte le procedure (programmazione, progettazione, appalto, esecuzione e collaudo), intanto iniziando a utilizzare quel lavoro che avevamo fatto nella legge semplificazioni, purtroppo fortemente Presidente, ho parlato di Sud: il 34 per cento è poco, perché significa soltanto continuare a dare quel che c'è già. Per ridurre il *gap* bisogna dare di più e diceva don Milani non c'è ingiustizia maggiore che fare parti uguali tra disuguali. Chiudo con la misurabilità. Dicevo che ci sarà un numero che ci giudicherà: se nel 2026 la somma degli investimenti pubblici in infrastrutture sarà *n* volte quanto investito nel 2019, con *n* sensibilmente maggiore di 1, avremmo trasformato l'Italia, reso migliore la vita degli italiani e fatto ripartire l'economia. Se quell'*n* non sarà maggiore di 1 questa generazione politica avrà perso la propria sfida, l'economia non ripartirà, l'Italia sarà nuovamente in ginocchio. Pertanto la misurabilità degli sforzi che faremo, a mio avviso, deve essere uno sprone per fare presto e bene, perché non ci saranno alibi.

sia il frutto di uno sforzo importante e ringrazio i Presidenti delle Commissioni e tutti i colleghi che vi hanno lavorato. Essa naturalmente sconta il passaggio tra il Governo Conte e il Governo Draghi. Io vorrei fare solo due considerazioni generali.

piano Marshall, un grande salto, che non è relativo solo alla vicenda della pandemia e alle conseguenze drammatiche della crisi economica. Per la verità, noi che siamo un Paese che, ancora prima della pandemia, non aveva recuperato il *gap* della crisi del 2008 e aveva problemi strutturali, di base produttiva, di produttività, di qualità ed efficienza dei servizi, siamo di fronte alla necessità di un cambio di paradigma. Io non so - lo dico con sincerità e onestà intellettuale - se effettivamente la classe dirigente di questo Paese

Si tratta di un vero e proprio salto e, quando fai un salto in una crisi, devi mettere in conto anche rotture, cambi radicali di direzione.

o è impensabile poter recuperare le grandi disuguaglianze che si stanno attraversando, sia territoriali, sia di genere, sia sociali. Questo cambio di prospettiva e di sviluppo richiede alcuni elementi e scelte radicali.

che promuova processi di sostegno all'accumulazione e la costruzione di nuove filiere produttive. Transizione ecologica non significa

facciamo come prima: no. Noi dobbiamo decidere come investire le risorse in politica industriale. Industria 4.0 investe su nuove filiere o diamo risorse a pioggia? Guardate, si tratta di una scelta difficile e, per alcuni versi, anche dolorosa. Transizione ecologica vuol dire stabilire i tempi per riconvertire un sistema industriale e contemporaneamente affrontare il tema del lavoro e la possibilità di sostituire un impianto industriale legato a un vecchio modello di sviluppo con nuove filiere industriali. Ora, io sono contentissimo del Ministero per la transizione ecologica, ma volete sapere quello che penso? Io penso che Mise, Transizione ecologica e Politiche agricole sono un unico progetto, che deve produrre un processo di trasformazione radicale. ma la devo dire lo stesso: noi siamo un Paese singolare. Negli Stati Uniti e in tante parti del mondo si discute della crisi del capitalismo, del fallimento di un'impostazione neoliberista e si cerca una nuova strada.

ma noi siamo di fronte al tema del lavoro dell'algoritmo e della frantumazione del lavoro. La prima questione che dobbiamo affrontare è riunificare il lavoro e trovare forme che rimettano insieme il lavoro. Questo è il primo punto: un grande cambiamento richiede una classe dirigente consapevole, che discute e si confronta, con una dialettica

i tempi, la trasparenza e la lotta alla criminalità organizzata. Attenzione a quello che sta succedendo e a quello che comincia a venire fuori

perché non c'è più la competenza. È una grande scelta di cambiamento, ci vuole coraggio. Concludo: non bastano i migliori, ma occorre la classe dirigente e la politica, quindi spetta a tutti noi.

sicuramente proficuo nelle Commissioni. Vorrei sottolineare alcuni aspetti. C'è un punto che credo sia noto a tutti noi; mi riferisco al fatto che il Governo e la maggioranza che lo sostiene convintamente nascono proprio dal fatto che, oltre all'emergenza pandemica, era necessario vedere, programmare, strutturare e - passatemi il termine - risistemare tutta quella che era la partita del *recovery* e, quindi, i piani che dovevano essere analizzati.

devono essere chiare per un motivo molto semplice. Sempre il Ministro ieri - spero voglia ribadirlo anche oggi - ha detto alla Camera

e i modelli organizzativi con riferimento ai presìdi sia per il coordinamento a livello centrale che a livello di enti. Tutto questo può far sì che tante cose siano lasciate fuori.

a livello centrale e deve essere partecipata. I relatori, con forme diverse, quando ieri hanno introdotto il loro ragionamento, hanno posto l'accento su questa

Italia. Spendo due parole su questo aspetto perché credo che il collega abbia voluto dire una cosa

C'è una fascia dell'Italia centrale che sta scivolando fondamentalmente verso il Sud per i parametri. Ritengo che alcune cose possano essere fatte sicuramente

Si sa benissimo, tanto per fare un esempio banale, che il Centro Italia svolterebbe se avesse l'Alta velocità, si sa benissimo quali sono i piani e i programmi. È quindi necessario stabilire inevitabilmente dei supporti che colmino questi *gap*, affinché non ci troviamo di fronte a

quella lista di 557 progetti che andavano dall'acquario *green* di Taranto a rifare il piazzale della Farnesina (permettetemi, la politica estera italiana non può certo passare dai 14 milioni di euro spesi per rifare i marmi di un piazzale). di strada ne abbiamo fatta. L'abbiamo fatta in maniera responsabile - e rispondo al collega Errani - cercando di essere classe dirigente e di governo di questo Paese. La cosa più importante

di scostamento in scostamento con il prossimo arriveremo ad impiegare una cifra addirittura superiore. Vorrei ricordare quegli scostamenti: 11 marzo 2020, 20 miliardi; 24 aprile 2020, 55 miliardi; 23 luglio 2020, 25 miliardi; 20 novembre 2020, 8 miliardi; 20 gennaio 2020, 32 miliardi. Il totale fa 140 miliardi ma, se aggiungiamo i 25 miliardi di *deficit* della manovra di bilancio, siamo a 165 miliardi. E il prossimo scostamento o i prossimi sicuramente ci porteranno a spendere di più. L'auspicio è di riuscire a farlo bene, perché non è che siano soldi gratis, ma soldi che i nostri figli dovranno ripagare. cento delle risorse previste andranno alla transizione ecologica. Permettetemi di soffermarmi su questo. Oramai è chiaro da dove partiamo e anche dove vogliamo arrivare. Ebbene, non ci si arriva coi monopattini elettrici prodotti in Cina. Questo è il problema più grande: superare un'impostazione sbagliata e ideologica, e andare a ragionare - questo abbiamo voluto fare - dei modi, dei tempi e dei costi e benefici dei singoli interventi, e soprattutto - permettetemelo - delle priorità, perché purtroppo non si può fare tutto. Uscire dalle ideologie significa anche - per citare il collega Margiotta - parlare sì dei porti al Sud e magari della Sicilia trasformata in un *hub* in mezzo al Mediterraneo, ma senza ponte sullo Stretto diventa un po' difficile; e non è che si possa pretendere di spostare Trieste o Genova e pensare che non arrivino lì determinate merci. Essere un Paese insieme non significa rivendicare - permettetemi di dirlo dal Centro - una questione meridionale a fronte dello sforzo che sta facendo il Nord, che è quello che ha subito di più la pandemia e che ha contato anche più morti; significa invece ragionare come un Paese unico. E farlo relativamente all'ambiente significa puntare sulla riduzione della dispersione idrica: l'acqua è un bene importante e non possiamo avere zone d'Italia in cui, per far arrivare un litro d'acqua in una casa, bisogna farne partire due, perché la metà si perde per strada. Significa che non si può avere in Sicilia l'80 per cento dei centri abitati privi di una depurazione funzionante. Questi sono gli investimenti da fare, perché permettono alle aziende di lavorare, investire, e dare risposte ai cittadini. Lo stesso vale per l'efficientamento energetico: i tre quarti degli edifici sono in fascia G,

che danno ricchezza, perché hanno una ricaduta importante anche sul turismo, perché il fatto che un terzo delle coste messinesi non siano balneabili è un danno non solo all'ambiente e alla salute, ma anche al turismo, come ricordava il ministro Garavaglia durante le audizioni in Commissione. Quindi, anche stabilizzare i livelli dei laghi italiani e puntare sulla qualità dell'ambiente significa tutelare e far prosperare il settore turistico. Questa Questa è l'impostazione che la Lega ha voluto inserire all'interno del PNRR. Un altro tema fondamentale è il ciclo dei rifiuti: è bello puntare a rifiuti zero, ma non lo si può fare senza impianti. La vergogna di avere 200.000 camion che spostano rifiuti dal Sud al Nord, dove si trovano deve finire. Con i fondi del *recovery* e gli altri che metteremo in campo potremo finalmente colmare questo divario. Tutto quello che viene utilizzato per la transizione ecologica non è un costo, è un investimento. Sta a noi far sì, un po' come nella parabola dei talenti, che da questo settore, permettendo alle imprese di investire e ai cittadini di vivere meglio, possano provenire le risorse per pagare il debito che stiamo contraendo. Lo dobbiamo non all'Europa, ma a noi stessi e ai nostri figli. *(Applausi)*.

una transizione necessaria per portare riequilibrio fra il sistema economico e quello sociale ed ambientale. L'economia ha il compito di migliorare la qualità della vita di una comunità, ma una comunità, a sua volta, ha il dovere di tutelare l'ecosistema, che è il macrosistema che contiene il tutto e senza il quale non potremmo più avere nessuna forma di economia, sia essa post-keynesiana, lineare, *green*, circolare, attenta all'ecologia profonda, all'ecologia integrale. Per noi del MoVimento 5 Stelle la parità di genere, l'attenzione ai nostri giovani e il rilancio del Sud sono obiettivi basilari. Non possiamo risollevare l'economia italiana se non colmiamo il divario fra i territori, se non aumentiamo la percentuale di donne in ambito lavorativo e se non le poniamo in ruoli decisionali, se non creiamo le condizioni per la creazione di posti di lavoro *green* per i nostri figli. In questo modo li richiamiamo dall'estero, perché delle loro menti brillanti, della loro creatività, dei loro sogni noi abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno per ricostruire un'Italia che sta resistendo con sacrificio e sta combattendo questa pandemia che accomuna tutti, ci pone tutti sullo stesso piano e ci fa capire come l'essere umano non può controllare tutto. Noi del MoVimento 5 Stelle siamo accanto ai cittadini da sempre. Siamo semplicemente i portavoce di chi ha bisogno, di chi lotta ogni giorno per poter aprire il proprio negozio, di chi è costretto a insegnare ai propri alunni stando dall'altra parte dello schermo. Che fine ha fatto la relazione? Purtroppo siamo costretti a questo per quello che ci sta accadendo.

di cui oggi stiamo discutendo in quest'Aula non sia *greenwashing.* *(Applausi)*. Occorre dunque evitare che vengano finanziati solo i progetti già pronti. Dobbiamo favorire una progettualità innovativa, altrimenti si rischia di avere un moltiplicatore di squilibri di genere, generazionali e territoriali. Qui non si tratta solo di valorizzare e investire nelle zone macroeconomiche speciali (ZES), oppure costruire infrastrutture, raccogliere, riusare e riciclare i rifiuti (quindi fare economia circolare), decarbonizzare (passando dall'energia fossile a quelle rinnovabili), diminuire gli sprechi di energia e risorse naturali, rendere la nostra agricoltura sostenibile. Sono tutte azioni validissime, ma c'è dell'altro. Oggi siamo chiamati ad affrontare l'era della resilienza e dell'antropocene e virare dall'antropocentrismo al biocentrismo. Io avrei dato un altro nome a questo piano, denominandolo piano nazionale per la cura della casa comune. È questo che i nostri giovani ci hanno chiesto nelle piazze: dateci un futuro, tutelate la nostra casa, salvate il nostro pianeta dai cambiamenti climatici che hanno già causato eventi dannosi, dal depauperamento del capitale naturale e dall'inquinamento. Dobbiamo proteggere, preservare e ripristinare la biodiversità, nonché i nostri mari, i fiumi, il suolo, i nostri paesaggi e l'aria che respiriamo. Dobbiamo tutelare la bellezza della nostra Italia, quella che tutti ci invidiano: sia quella naturale, che quella costruita dall'uomo, con le nostre bellezze culturali. Dobbiamo attuare l'Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU. Dobbiamo dare un vero impulso al *Green Deal* europeo, misurare la sostenibilità per tutelare l'ambiente e attuare una giusta ripresa economica, utilizzando dei metodi come la valutazione del ciclo di vita e indicatori come la *carbon footprint* per certificare processi e tecnologie e creare un mercato di servizi e prodotti ecosostenibili. È necessario, ad esempio, tutelare le api per il loro servizio ecosistemico che tutti dimentichiamo. incentivare l'utilizzo di refrigeranti naturali per la catena del freddo, per eliminare i gas fluorurati fortemente impattanti per il cambiamento climatico, ma ancora molto utilizzati in Italia. Dal *blog* di un caro amico che stimo: sono trent'anni che parlo, grido e scrivo della tutela dell'ambiente, del contrasto al consumismo, della riduzione dell'uso di energia, dei materiali e del tempo di lavoro. In buona parte, grazie al MoVimento 5 Stelle, grazie al MoVimento 5 Stelle, questi temi sono finalmente arrivati in Parlamento e poi al Governo. anni dalla fondazione del MoVimento 5 Stelle, il 4 ottobre 2009, giorno di san Francesco, molti dei nostri obiettivi fanno parte dell'agenda di Governo di un Paese del G7, la nostra Italia. Il MoVimento 5 Stelle è nato per portare al Governo le migliori idee innovative per la tutela della nostra casa comune e per creare lavoro utile e rendere competitivi in un mercato sempre più *green* le nostre filiere produttive. Per questo ha chiesto l'istituzione del Ministero per la transizione ecologica (MiTE). Come sarà il mondo dopo quello che ci sta accadendo? Sta a noi decidere. Se vogliamo che sia migliore nessuno deve essere lasciato indietro. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza non può fallire. Servono una *governance* efficace, il coinvolgimento del Parlamento, un giusto processo riformatore, una visione sistemica biosferica e un nuovo approccio culturale. È un approccio che il MoVimento 5 Stelle ha sempre portato avanti. Noi ci saremo e continueremo a farlo.

abbiamo fatto un immane lavoro di ascolto e di sintesi di contenuti importanti, che credo possano colmare alcune lacune evidenti,

tempistica e i progetti. Signor Ministro, dobbiamo fare in modo che si scongiuri il rischio che, in nome di questa tempistica stringente e dei criteri altrettanto esigenti che il Piano ci chiede, vengano finanziati solo i progetti oggi già pronti. Rischieremmo di mettere dentro progetti vetusti, che stanno nei cassetti dei Ministeri da anni, ma soprattutto temo che questo principio, in pratica, si possa tradurre nell'allargare il divario che esiste tra i territori. infatti del tutto evidente che i territori che si misurano con qualche difficoltà in più, hanno qualche problema in più, anche strutturale, da risolvere. Quindi, credo che dobbiamo trovare un equilibrio rispetto a questi temi. altro tema che voglio mettere in evidenza anche qui, oggi, e lo dico senza aver paura di farlo con il titolo giusto: il Mezzogiorno. Il Piano ha una dotazione finanziaria così elevata perché, in virtù dei tre criteri che l'Europa ha voluto analizzare, ha rilevato, soprattutto nella parte a Sud del Paese, dei *deficit* infrastrutturali importanti, ma anche dei *deficit* economici importanti. Popolazione residente, PIL *pro capite* e occupazione sono gli indici che hanno fatto sì che l'Europa ci destinasse il 25 per cento della dotazione complessiva. Stiamo attenti:

metà. Credo che l'Alta velocità debba essere un diritto universale, al Sud come al Nord, perché non è possibile avere due Paesi in uno. Infine, riallocazione delle risorse liberate, sappiamo che il Piano libera risorse, perché progetti che erano già stati finanziati in questo Piano trovano posto e quindi liberano risorse. Attenzione a mettere quelle risorse risorse sui progetti che non hanno i requisiti stringenti del regolamento 2021/241, ma che hanno un interesse nazionale. Penso - lo ripeto - all'Alta velocità, ma anche all'ammodernamento della rete stradale e autostradale, anche al Sud.

Ci vuole trasparenza, legalità, affermazione dei princìpi costituzionali, ma ci vogliono delle procedure *ad hoc,* altrimenti non si il ruolo del Parlamento e credo, signor Ministro, che in questo ci deve aiutare. Dobbiamo avere infatti un ruolo di interlocuzione. Vogliamo con forza che queste indicazioni vadano nella bozza definitiva del PNRR, ma vogliamo soprattutto che il Parlamento continui a restare informato sull'evoluzione, attraverso delle valutazioni periodiche nelle Commissioni che si sono occupate del PNRR, che credo contribuiranno che credo contribuiranno anche a rafforzare l'azione del Governo. Signor Ministro, conosco la sua sensibilità e spero che il Parlamento possa venire a conoscenza dei progetti reali.

È stato anche necessario fare questa operazione di ascolto del sistema Italia, che non si era fatta che costituiva un altro limite. Noi l'abbiamo fatto: abbiamo ascoltato circa 300 soggetti. È stato utile e credo che la relazione sia un'ottima sintesi delle aspettative del Paese. Le rinnovo l'invito a interloquire con noi con la stessa disponibilità manifestata fino a questo momento. Ringrazio anche il Sottosegretario e, soprattutto, i colleghi della 14a e 5a Commissione per il lavoro condiviso.

Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Sartore per essere stata qui per tutta la discussione e il Ministro per aver partecipato questa mattina alla discussione. Penso sia un fatto importante che anche lei possa prendere coscienza direttamente delle

Parto dalla sanità. Sono intervenuti i colleghi Giuseppe Pisani e Mautone, ma anche una collega della Lega che ci ha fatto capire quali sono le vere difficoltà che sta vivendo oggi il settore della sanità con riferimento proprio anche al personale che manca, al personale necessario soprattutto

necessario investire nel turismo, nelle aziende creative e in quelle che producono contenuti di spettacolo per fare in modo che il nostro Paese si possa riprendere in un campo in cui siamo sempre stati maestri e dobbiamo continuare a esserlo. Per farlo bisogna investire nelle strutture. Abbiamo lo strumento del superbonus; dovremmo riuscire

ci ha fatto capire quanto sia importante, parlando di pubblica amministrazione, investire nelle competenze. Purtroppo, siamo in un periodo, che dura da molti anni, nel quale sono state rinnovate poco le risorse umane all'interno dei Comuni e degli enti territoriali.

questo immenso progetto che mira a far ripartire la nostra nazione. Ricordo ancora tutti i colleghi che hanno parlato di ambiente. Sull'ambiente mi soffermerei in modo particolare, Ministro. Come ho ricordato ieri - lo ricordo ancora oggi e l'ho ricordato anche il 13 ottobre quando abbiamo presentato la nostra relazione sulle linee guida vi è un'assenza forte in questo progetto, che è la tutela degli ecosistemi, la tutela degli ambienti marini, costieri, del territorio. Purtroppo, in Italia abbiamo patito per decenni veri drammi ambientali cui è necessario porre riparo. So che servono risorse straordinarie; so anche, però, che laddove si sono verificati danni, si possono andare a trovare le risorse da chi quei danni li ha creati. Non è facile, ma dobbiamo impegnarci. che parla di rinascita, ripresa, rilancio, partendo dall'ambiente, deve per forza impegnarsi un po' di più sull'ambiente, e quindi trovare il modo di riuscire a ripristinare laddove i danni sono stati creati; ripartire dalle infrastrutture verdi, dalle aree naturali che servono e che forniscono servizi ai cittadini.

quell'aspetto di *greenwashing* che ci hanno ricordato i colleghi Pellegrini, L'Abbate, ma anche molti altri, per quanto riguarda il fatto che alcuni investimenti sembrano verdi, ma in realtà poi tali non sono perché il loro impatto sull'ambiente può essere veramente distruttivo. Bisogna fare in modo che le risorse vengano spese bene. Mi ricollego a quanto detto prima dal collega Stefano; ribadisco anche io la mia richiesta. Anzitutto, Ministro, ci serve capire come questo Piano arriverà in Parlamento, non dico per essere approvato ma quantomeno per dare contezza al Parlamento e quindi al Paese dei contenuti reali che state mettendo a punto in questi giorni.

noi abbiamo analizzato un documento che comunque è il Piano su cui state lavorando, un piano un po' vecchio. Ci servirebbe sapere invece quali sono le modifiche che state apportando. La collega Gallone ha assicurato che il Piano è totalmente rivoluzionato;

quindi, vi chiedo quali siano gli aspetti innovativi che state aggiungendo perché per noi è fondamentale saperlo per dare risposte anche ai cittadini. Ministro, le faccio questa preghiera: ci mandi prima possibile degli elementi per fare in modo che i nostri cittadini sappiano quali sono i veri contenuti di questo Piano.

finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, anzitutto vi ringrazio per l'invito a replicare in alla discussione della relazione delle Commissioni riunite sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza. resilienza. Vi ringrazio anche per le molteplici indicazioni fornite nei vostri interventi sia ieri sia questa mattina; sono estremamente costruttive e preziose per il seguito del nostro lavoro. Mi dispiace e mi scuso di non essere stato qui ieri all'avvio dei vostri lavori in relazione all'attività del Consiglio dei Ministri. Come ho già sottolineato nella mia audizione presso le Commissioni congiunte l'8 marzo scorso, il Piano nazionale è una grande occasione per avviare un processo di crescita duratura per il Paese, che esce da circa un quarto di secolo di crescita piuttosto scarsa o comunque modesta rispetto agli altri principali Paesi europei. La buona riuscita del Piano richiede uno sforzo corale delle diverse istituzioni coinvolte e un dialogo aperto e costruttivo; richiede una strategia del Paese, una visione per quello che sarà il Paese nel 2026, nel 2030 e possibilmente nei decenni successivi. Parlamento delle note tecniche relative alle missioni componenti della prima bozza del PNRR, predisposta dal precedente Esecutivo e da cui è partito il nostro lavoro, partito il nostro lavoro, è stata guidata dalla volontà di facilitare un dialogo stretto tra Parlamento e Governo, nell'ottica della più completa trasparenza. La bozza del Piano su cui stiamo lavorando ha un contenuto informativo che diventa via via più ricco, ricco, in coerenza con i requisiti europei ma anche e soprattutto per consentire una valutazione approfondita da parte delle istituzioni e dell'opinione pubblica. Ogni euro che verrà impegnato, ogni euro che verrà speso dovrà essere rendicontato. Ricordo che anche i contributi a fondo perduto impongono un onere per il bilancio europeo a cui il nostro Paese è poi tenuto a contribuire. Il Parlamento in questi mesi ha svolto un prezioso lavoro di interlocuzione con istituzioni e parti sociali. Il lavoro svolto dalle Commissioni riunite bilancio e politiche dell'Unione europea, congiuntamente alle altre Commissioni permanenti nei diversi ambiti di competenza, è stato serrato e impegnativo. Sono state raccolte le osservazioni e le istanze di numerosissimi soggetti (istituzioni, associazioni di categoria, esperti); come è stato appena detto, si è trattato di un grande esercizio di ascolto della società italiana. Il lavoro di sintesi del Parlamento, che confluisce nelle relazioni delle Commissioni sul Piano nazionale e nelle risoluzioni votate dal Senato e dalla Camera, contribuirà decisamente alla fase finale di definizione del Piano di qui alla fine del mese di aprile. È un lavoro ricognitivo molto approfondito che va pienamente utilizzato. L'impegno del Governo di avvalersi delle indicazioni contenute nelle risoluzioni, nelle relative relazioni, nella redazione della nuova versione del Piano e l'impegno di coinvolgere il Parlamento prima della sua trasmissione alla Commissione europea non discende solo da mero obbligo di ottemperanza nei confronti delle risoluzioni, ma anche e soprattutto dal convincimento che una condivisione strategica del Piano sia possibile soltanto attraverso il pieno coinvolgimento di tutte le istituzioni, in primo luogo del Parlamento. Questo, ovviamente, non riguarda soltanto la fase di predisposizione attuale, ma anche tutta la successiva fase di attuazione fino al 2026. Alla luce delle osservazioni, delle relazioni e degli interventi odierni in Aula, permettetemi di condividere con voi qualche considerazione circa l'attività che stiamo svolgendo in queste settimane. Come sapete, il coordinamento di quest'attività è incardinato al Ministero dell'economia e delle finanze. Ci tengo però a dire che tutto il Governo è coinvolto nella redazione del Piano. Come sapete, la Commissione europea ha definito, attraverso le sue linee guida, i piani di ripresa e resilienza come piani che devono essere di riforma e di investimento. L'accento sulle riforme è fondamentale, non solo per garantire l'efficacia e la rapida attuazione degli stessi investimenti, ma anche per superare quei nodi strutturali che hanno per lungo tempo determinato nel nostro Paese una crescita insoddisfacente e livelli occupazionali inadeguati soprattutto per i giovani e per le donne. Molti di questi punti di debolezza sono stati ricordati questa mattina. Si è ricordato anche, per esempio, come la lista delle questioni da affrontare ora vada in realtà indietro nel tempo. La dotazione di risorse per l'Italia del fondo di ripresa e resilienza è stimata pari complessivamente a 191,5 miliardi di euro; di queste risorse circa il 60 per cento dovrà essere destinato a obiettivi di modernizzazione digitale del Paese e di transizione ecologica, con particolare riferimento alla lotta al cambiamento climatico. Sono criteri precisi, rilevanti e impegnativi. Non sono solo la chiave per costruire un'Italia più moderna e più verde. Sono anche obiettivi indispensabili per rimanere al passo con lo sviluppo europeo, creando un ampio mercato per prodotti, servizi e nuove competenze, dal quale le nostre imprese e i nostri giovani potranno trarre pieno vantaggio. Dobbiamo far sì, con questo Piano, che i giovani e le imprese siano al centro del nostro sforzo di ripresa. Mi riferisco, qui, alle imprese di tutti i settori: innanzitutto, il settore manifatturiero; i servizi, tra i quali, ovviamente, è fondamentale il turismo; l'agricoltura, che è stata spesso ricordata questa mattina. Il Piano deve aiutare la trasformazione e il rafforzamento del nostro sistema produttivo. Tengo a ribadire, come ho già evidenziato in altre occasioni, che il Piano è un'occasione di sviluppo molto importante per il nostro Paese, ma non è l'unico strumento di politica economica per raggiungere obiettivi di crescita, inclusione ed efficienza. La strategia di politica economica deve includere i fondi strutturali europei, il fondo di sviluppo e coesione, oltre che, naturalmente, la legislazione ordinaria. Ricordo che i fondi di investimento di durata di 15 anni, inclusi nelle ultime cinque leggi di bilancio, prevedono investimenti per quasi 200 miliardi. Questo mi conduce a due osservazioni. La prima è che il Piano è uno strumento aggiuntivo prezioso. A questo proposito, vorrei dire che una parte significativa dei progetti finanziati con il PNRR riguarderà iniziative nuove. Inoltre, preciso che l'individuazione e la definizione, sia dei progetti in essere sia dei nuovi progetti, si basa su criteri volti a concentrare le risorse sugli interventi più innovativi, a maggior impatto sull'economia e sul lavoro. Occorrerà evitare che la spesa aggiuntiva per investimenti prevista dal Piano sia compensata da una minore spesa ordinaria, come accaduto in altri casi in passato. Per questo, dobbiamo migliorare la nostra capacità di gestire progetti di investimento, il che richiede procedure più efficaci e snelle (questo punto è stato ricordato molto spesso questa mattina) e anche strutture tecniche, nelle pubbliche amministrazioni, centrali e non centrali, che siano più solide. Seconda osservazione. È importante rammentare che i progetti che non fossero inclusi nel Piano non saranno necessariamente accantonati. Non solo esistono gli altri strumenti nazionali ed europei, ai quali facevo cenno in precedenza, ma stiamo pensando anche a costituire una linea di finanziamento *ad hoc*, complementare al Piano, che includa i progetti di investimento che, pur meritevoli di essere inclusi nel Piano per spirito e finalità, ne siano esclusi perché non soddisfano alcuni criteri più stringenti. Vorrei anche soffermarmi su come la predisposizione del Piano, che ci vede impegnati in questi giorni, stia incorporando i tre temi trasversali riguardanti l'inclusione che il Piano si prefigge di affrontare: la parità di genere, i giovani e gli squilibri territoriali. L'intero Piano è improntato a una prospettiva di riequilibrio dei differenziali di genere e include misure volte a garantire una parità sostanziale nei diversi ambiti, non solo lavorativo, ma anche sociale e culturale. In questo quadro, il Piano prevede azioni di sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità femminile e l'attuazione di diversi interventi abilitanti, a partire da un deciso rafforzamento dei servizi sociali, quali gli asili nido. Inoltre, l'obiettivo di garantire la piena partecipazione dei giovani alla vita culturale, economica e sociale del Paese, investendo in istruzione e ricerca e intervenendo con politiche per incrementare il livello di occupazione giovanile, nel breve e nel lungo periodo, è trasversale a tutto il Piano. Al di là degli effetti indiretti a favore dei giovani, derivanti dallo sviluppo dei nuovi settori perseguito dal Piano, si prevedono impatti diretti sulle nuove generazioni, in particolare nella missione istruzione e ricerca, con progetti dedicati al contrasto dell'abbandono scolastico, alla digitalizzazione della didattica, al potenziamento della ricerca; e nella missione inclusione e coesione, con interventi sulle politiche attive e sul lavoro e il potenziamento del servizio civile universale. Scuola, università, capitale umano sono cruciali per il nostro Paese. Dobbiamo anche superare le cicatrici indotte dalla pandemia sui processi di apprendimento l'anno scorso e quest'anno. Uno degli elementi centrali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, vale a dire la decisa trasformazione della nostra economia verso un paradigma di crescita inclusiva e sostenibile, costituisce di per sé un grande contributo al benessere e alla qualità della vita delle giovani generazioni. Ricordo che la questione climatica è anche una delle priorità della Presidenza italiana del G20. G20. Il Piano nazionale contribuirà a ridurre gli squilibri territoriali. Anche in questo caso opererà con due modalità: una diretta, attraverso il finanziamento di interventi localizzati nel Mezzogiorno, e una indiretta, attraverso azioni di carattere trasversale che hanno un forte impatto sulle aree del Sud e delle Isole. Nel complesso, le risorse destinate alle aree territoriali del Mezzogiorno supereranno significativamente la quota del 34

ricordato questa mattina), la scuola, la sanità, l'agricoltura, gli asili nido ed altri comparti. La debolezza economica del Meridione ha cause complesse che richiedono un'azione su più fronti. Un ultimo aspetto su cui vorrei soffermarmi riguarda la *governance* del Piano, in particolare relativamente all'interlocuzione tra Governo centrale ed enti territoriali. Come giustamente sottolineato nelle relazioni del Senato e della Camera, la definizione di una *governance* snella e ben definita a livello centrale delle autonomie territoriali è senz'altro un nodo cruciale. Nel raccogliere la sollecitazione del Parlamento su questo punto, vi anticipo che la proposta finale di Piano conterrà la descrizione di un modello organizzativo basato su una struttura di coordinamento centrale, collegata a specifici presidi settoriali preso tutte le amministrazioni coinvolte, unitamente a strumenti e strutture di valutazione, sorveglianza e attuazione degli interventi. Questa cornice assicurerà una sana gestione finanziaria, il rispetto delle regole europee e nazionali e il rispetto degli obiettivi quantitativi e dei traguardi intermedi. Inoltre, al fine di facilitare un'efficace e tempestiva attuazione del Piano, è prevista la definizione di un pacchetto di norme di semplificazione procedurale che agevoli la concreta messa in opera degli interventi, anche nel caso di interventi la cui realizzazione sarà responsabilità degli enti territoriali. La questione delle procedure, come spesso ho ricordato questa mattina, è la sfida più importante con cui dobbiamo confrontarci. Su questo punto, come su quello delle riforme, che è fondamentale nella costruzione di un Piano efficace, il Parlamento avrà un ruolo centrale nell'assicurare un contributo significativo o un dibattito ampio, ma anche una concreta capacità di individuare in tempi rapidi le soluzioni più opportune nei vari passaggi parlamentari, richiesti nei prossimi mesi ed anni per la realizzazione delle riforme. Infine, la *governance* prevista assicurerà adeguate modalità di aggiornamento del Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi e sul raggiungimento degli obiettivi. In particolare, sarà resa disponibile una piattaforma digitale pubblica centralizzata con i dati relativi all'attuazione dei progetti del Piano. In conclusione, il Piano rappresenta una sfida organizzativa complessa, soprattutto - torno a dire - nella fase di attuazione. Esige una visione strategica e una capacità progettuale ed attuativa che stiamo cercando di calare nel Piano stesso. Dobbiamo completarlo e farne uno strumento di sviluppo e ridisegno del Paese. In questo ci aiuteranno le risoluzioni approvate dal Parlamento. *(Applausi)*.

«impegna il Governo a trasmettere al Senato, con cadenza periodica, in relazione alle scadenze europee, la necessaria documentazione relativa al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da consentire alle Camere di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto dei tempi e degli obblighi di risultato previsti dal regolamento UE/2021/241».

Con la votazione degli atti di indirizzo si intende esaurita la discussione del Documento all'ordine del giorno.

Presidente, signori Ministri e Sottosegretari, colleghe e colleghi, nonostante i tempi ristretti, le Commissioni sono riuscite a elaborare una serie di riflessioni che arricchiscono il percorso per la redazione definitiva del Piano una mole di considerazioni su cui è impossibile dar conto in pochi minuti. Forse sarebbe stato meglio un documento più agile, che indicasse la *governance* e la strategia sulle riforme, senza entrare nel dettaglio della progettualità. Mi limiterò quindi ad alcuni punti, ma, se c'è un concetto fondamentale espresso nella relazione, è quello del diritto alla ripartenza delle imprese. Dopo tredici mesi di rallentamenti e chiusure, gli aiuti da soli non bastano, ma devono innestarsi su un contesto radicalmente diverso. Il primo punto del nuovo contesto riguarda il ruolo degli istituti di credito. Com'è scritto nella relazione, le attuali norme bancarie rischiano di tramutarsi in un ostacolo per l'accesso al credito da parte delle aziende che hanno tutte le carte in regola per rilanciarsi sul mercato e che scontano solo un problema di liquidità. È un aspetto che andrà osservato con grande attenzione, così come l'impegno per far sì che le riforme portino davvero a una maggiore efficienza del sistema. Bene allora le nuove assunzioni nella pubblica amministrazione, con l'obiettivo di immettere forze giovani e motivate competenze, che oggi mancano e che invece saranno decisive per lo sviluppo dei progetti. Bene l'impegno a una radicale semplificazione normativa, per fare in modo che l'Italia non venga ricordata come il Paese dove, per fare un'opera pubblica di 25 miliardi (che è il taglio medio dei progetti del *recovery*), ci vogliono non meno di dieci anni o dove, per aprire una gelateria, servono 73 adempimenti presso 26 enti e 13.000 euro. All'estero invece la certezza dei tempi è dettata dal meccanismo del silenzio-assenso e dal fatto che i controlli sono sempre *ex post*. Per questo occorrono subito la sospensione del codice degli appalti e una normativa che si limiti a recepire le linee essenziali richieste dall'Unione europea; subito occorre un taglio netto a quei colli di bottiglia burocratici che, come ci ricorda l'Europa, rischiano di vanificare anche una misura strategica quale quella del 110 per cento. Ha pertanto ragione il ministro Giovannini quando dice che, per l'avvio dei progetti infrastrutturali, non si deve aspettare il giudizio finale della Commissione europea.

4,5 miliardi per il *cashback* sono davvero troppi; risorse che appartengono alla collettività vengono riallocate tra chi ha maggiore capacità di spesa e questa distorsione su importi così ingenti è inaccettabile. Recuperiamo queste risorse per destinarle ad altri interventi, ad esempio per consolidare l'alternanza scuola-lavoro o per rafforzare le politiche abitative, su cui, nella relazione delle Commissioni, vengono spesi passaggi molto interessanti. Da un lato, si devono rafforzare gli strumenti per la sostenibilità dei mutui, ma, dall'altro, si deve anche guardare a quello che fanno gli altri Paesi, dove nei primi anni della nuova famiglia si paga solo la quota interessi e non la quota capitale. Un capitolo altrettanto importante è quello della riforma fiscale: non solo riduzione degli adempimenti e tassazione per i giganti del *web*, ma soprattutto un fisco al servizio della ripresa economica, con strumenti più efficaci sulla cessione dei crediti fiscali, cosa quanto mai necessaria per valorizzare le varie misure sulla riqualificazione del patrimonio immobiliare. Tra questo patrimonio devono rientrare anche gli alberghi e le strutture ricettive: il turismo dev'essere al centro del *recovery*, perché, come ha spiegato il professor De Rita, la ripresa passerà in gran parte da quei settori che hanno una capacità di trascinamento per l'intera economia e, tra questi, il turismo è il principale. Pertanto occorre non solo un sostanzioso rafforzamento delle misure del decreto sostegni, ma anche, come ha detto il ministro Garavaglia, l'ampliamento del superbonus del 110 per cento per finanziare l'antincendio e altri interventi che non riguardino solo l'efficientamento energetico. Altro tema è la montagna. La pandemia ha aumentato le difficoltà dei nostri territori. Per questo, quando si parla di riduzione dei divari territoriali, non lo si deve intendere solo come quello tra Nord e Sud, ma anche come quello tra piccoli e grandi centri, tra realtà interne e costiere, tra pianura e montagna. Nel testo che oggi approviamo c'è un impegno molto forte alla digitalizzazione e questo è sicuramente uno dei nodi più importanti, dato che, solo per fare un esempio, tra le aziende agricole solo il 4 per cento è digitalizzato. Crediamo però che non basti: serve una riflessione di sistema su come declinare i grandi obiettivi del Piano rispetto alla specificità di questi territori. Dalla lotta allo spopolamento a quella contro il dissesto idrogeologico, dalla tutela della biodiversità alla salvaguardia delle attività economiche, dalla questione generazionale all'agricoltura, la montagna richiede interventi calibrati. Concludo, signor Presidente, con alcune riflessioni sulla *governance*. La prima è che non è ancora chiara l'architettura e in particolare chi svolgerà il ruolo di stazione appaltante, che non è di certo un aspetto secondario sulla possibilità di riuscita del Piano. Credo che questo nodo vada sciolto quanto prima, attribuendo un ruolo centrale alle Province, che saranno importanti soprattutto nei territori in cui non ci sono grandi realtà amministrative. riflessione riguarda la definizione di un criterio per stabilire quali progetti saranno finanziati con i contributi a fondo perduto e quali mediante prestiti, come pure la specifica sezione per i progetti che per motivi di tempo o di cantierabilità rimangono formalmente fuori, ma che possono essere recuperati con i fondi ordinari della programmazione europea. Importantissimo sarà anche il ruolo del Parlamento sul monitoraggio e sul controllo dello stato di avanzamento dei progetti con criteri quantitativi e qualitativi, oltre che naturalmente in tutti i passaggi che ci attendono in questo mese. Ancora più importante sarà però la discussione che nei prossimi mesi nascerà in Europa. Dobbiamo fare in modo che il *recovery plan* diventi un elemento strutturale della politica europea per accelerare così il processo di integrazione. Questa crisi ci ha ricordato l'importanza e il valore assoluto dell'Europa. L'Italia ne uscirà, se saprà davvero vivere le prossime settimane con coraggio e radicalità delle scelte. Il *recovery* è un'opportunità storica: sfruttiamola fino in fondo.

oggi che continuiamo a piangere i nostri morti e a valutare il costo economico e sociale della pandemia, di fronte alla speranza di una non lontana via d'uscita rappresentata dai vaccini, per i quali abbiamo finalmente un piano, ci sentiamo meno fragili e meno vulnerabili. Ora non possiamo fallire la sfida che avevamo e che abbiamo ancora di fronte: riscrivere un nuovo Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo oggi è il nostro compito. La risposta europea, come abbiamo detto, c'è stata; dalla sospensione delle procedure del patto di stabilità, prorogata al 2023, sulle cui necessarie modifiche dovremo comunque riflettere presto,

Ora è il tempo della risposta nazionale che consenta di liberare tutto il potenziale di crescita, aggredendo con coraggio i punti di debolezza del sistema a partire dai bassi livelli di crescita annuale, la progressiva diminuzione demografica a cui il *family act* e l'assegno unico, approvato due giorni dare una risposta concreta a partire dagli alti livelli di disoccupazione e i bassi livelli di scolarizzazione. È proprio guardando al futuro che oggi siamo chiamati a pianificare le risorse a nostra disposizione del Next generation EU. È una grande responsabilità per noi che siamo uno uno dei maggiori beneficiari, con 209 miliardi, per affrontare certamente le attuali difficoltà generate dalla crisi, ma anche per il superamento delle persistenti divergenze territoriali tra un Nord e un Sud ancora troppo lontani, tra il centro e la periferia, per la lotta alle disuguaglianze sociali, ma anche generazionali e di genere. Sono risorse che dovranno accompagnare soprattutto la transizione ecologica - a cui destinare, signor Ministro, più del 37 compresa la biodiversità, obiettivo assente nel piano precedente - verso la neutralità climatica al 2050, ma anche la digitalizzazione, per uno sviluppo che dovrebbe essere duraturo, oltre che sostenibile, anche dal punto finanziario, per quel debito che abbiamo oggi, ma soprattutto per quello che dovranno ripagare i nostri figli. La relazione presentata oggi è importante e rende conto dell'utile lavoro portato avanti in questi due mesi dalle Commissioni riunite, con audizioni di portatori di interessi diffusi, enti locali e società civile, nonché le priorità indicate dai Ministri maggiormente coinvolti dal nuovo Governo. Di certo, il nuovo Piano deve tener conto delle indicazioni contenute nelle nuove linee guida della Commissione e soprattutto deve ancorarsi alle condizionalità previste dal recente regolamento del 18 febbraio. Occorre dunque riscrivere le sei missioni le misure che dovranno rispondere a principi generali importanti, a partire dalla parità di genere, ma anche a principi orizzontali quali l'addizionalità delle risorse - come lei, signor poc'anzi - il che implica che non potranno essere finanziate misure già contenute nel bilancio corrente o voci di spesa già coperte da altre risorse. condizionalità rispetto anche agli equilibri di bilancio. Il Piano sarà valutato in base alla coerenza, all'efficienza della spesa e alla pertinenza e dunque sarà in discontinuità con quello approvato dal precedente Governo Conte, che ci era invece apparso da subito carente sia in strategia sia in anima politica. Avevamo chiesto di fare in fretta e che vi fossero investimenti in opere e infrastrutture, nonché maggiori risorse per la sanità per i giovani, ai quali dobbiamo dedicare uno specifico pilastro, perché non basta considerarli come priorità trasversale o destinatari dell'intero Piano. Ripeto che occorre un pilastro specifico. Avevamo chiesto anche più risorse per la cultura e il turismo. un Piano che indichi finalmente una sana *governance*. Ritengo positivo concentrarla, signor Ministro, presso il suo Ministero in coordinamento con gli altri singoli Dicasteri e con gli enti locali. Questa per il nostro Paese è la grande sfida: superare i colli di bottiglia e i nodi strutturali che da sempre hanno rallentato la realizzazione di opere e un pieno ed efficiente impiego delle risorse europee verso procedure semplificate, con un maggior potere decisionale, anche anche sostitutivo, rispetto all'inerzia dei diversi soggetti attuatori, indicando altresì le modalità di controllo antifrode (come ci richiede la Commissione), con un monitoraggio costante dei risultati. Si tratta di condizionalità vere e proprie, dunque, il che significa che, accanto agli investimenti, dovremo avere la forza di realizzare le importanti riforme, indicate anche nelle raccomandazioni per Paese, del semestre europeo. Per noi significa soprattutto riforma della pubblica amministrazione, più semplice e più snella, anche con l'immissione di nuove competenze, per una cultura amministrativa finalmente orientata al risultato; riforma della giustizia, più efficiente, e riforma dell'istruzione, per il più importante dei fattori, ossia i nostri figli e la loro conoscenza, senza dimenticare la sanità

dipenda dal rafforzamento del mercato interno per riportare all'interno dell'area europea riascoltare strategiche di sicurezza, quali quelle sanitarie, a partire proprio dai vaccini. Next generation EU e la svolta europea, pur nell'incertezza delle ratifiche delle decisioni sulle risorse proprie, ma di certo il Piano nazionale di ripresa richiede la svolta italiana. Auspichiamo che il Piano possa contenere importanti previsioni, che indichiamo come priorità: transizione 4.0 per l'innovazione tecnologica delle imprese; connessioni veloci e intermodali (ferrovie e aeroporti, a partire dal Sud); trasporto pubblico locale verso la mobilità sostenibile; risanamento di edifici scolastici; più asili nido; interventi di efficientamento energetico; nuove fonti quali l'idrogeno, ma anche contrasto al dissesto idrogeologico; rigenerazione urbana e *housing* sociale. senza dimenticare, come dicevo prima, interventi per la biodiversità, di cui le acque interne sono preziose custodi. Signor Presidente, come ha suggerito, riconsideriamo la previsione contenuta nella precedente bozza del Piano, i miliardi per progetti in essere, perché non dobbiamo pensare solo di abbattere il debito pubblico che abbiamo oggi, ma piuttosto di renderlo sostenibile per il futuro, sprigionando una grande forza per il potenziale di crescita duratura. Inoltre, concordiamo con lei sulla non opportunità di inserire nel Piano la quota di risorse del Fondo di sviluppo e coesione (i famosi 20 miliardi previsti nel precedente Piano), che potremmo, al contrario, liberare dalle condizionalità di tempo e di procedure previste dal *recovery facility* per tenerle fuori, come riserva di interventi mirati al perseguimento dei medesimi obiettivi di coesione. Dunque, il PNRR è un autentico esame di maturità per il nostro Paese. Next generation EU è stato un passo decisivo verso un'Europa più integrata, con un debito comune, e un bilancio autenticamente europeo. Ora tocca a noi dimostrare di esserne all'altezza, perché, come ha detto il presidente Draghi in quest'Aula il giorno della fiducia, non c'è Europa senza Italia e fuori dall'Europa c'è meno Italia. Non manchiamo dunque l'opportunità che abbiamo di fronte. Abbiamo fiducia in questo Governo, quindi in attesa di un confronto qui in Parlamento con il nuovo PNRR, dichiariamo il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-P.S.I. alla proposta di risoluzione di maggioranza.

ed auspico che nelle sue repliche possa dare conferma rispetto ai temi che porremo e su cui non abbiamo ancora chiarezza, anche se, in qualche modo, è già intervenuto. Capirà a cosa mi riferisco, perché, come forse sa, signor Ministro, abbiamo depositato oggi una doppia risoluzione, cosa che di solito non accade, perché i Gruppi parlamentari

per quanto riguarda l'approvazione definitiva del Piano di ripresa e di resilienza, sul merito del quale si sono già espressi nel corso dei loro interventi i colleghi di Fratelli d'Italia, che ringrazio tutti, approfondendo molti dei temi che sono chiaramente di loro competenza.

la versione definitiva del *recovery plan*, che, come lei sa meglio di me, sarà presentato a Bruxelles il prossimo 30 aprile, ma anche eventualmente di incidere su questa proposta

È questo il motivo per cui il Gruppo Fratelli Italia ha chiesto che questo Piano possa seguire un percorso che assicuri la certezza dell'*iter* parlamentare evidentemente previsto dai Regolamenti di Camera e Senato, Senato, per dare certezza e garanzia di partecipazione al dibattito politico e a tutte le forze politiche presenti in questo Parlamento, compresa la forza politica che rappresento e che - lo voglio ricordare - è l'unico Gruppo parlamentare presente in quest'Aula all'opposizione di questo Governo.

Signor Presidente, troviamo di una gravità inaudita che il Parlamento non possa intervenire sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, che decide non solo gli investimenti dei prossimi anni, ma anche il futuro della Nazione nei prossimi decenni. Spero che il Ministro mi possa ascoltare, perché siamo l'unica forza di opposizione. Signor Ministro,

ingannare il Parlamento per quello che il Presidente del Consiglio dei ministri ci ha detto al momento del suo insediamento. Secondo noi sta venendo meno l'impegno chiaro di mettere al centro dell'azione politica il ruolo delle Commissioni e delle Assemblee parlamentari. Voglio ricordare anche che sul PNRR si è avuta una crisi di Governo - l'ennesima - e si sono svolti giochi di palazzo che hanno tenuto l'Italia paralizzata per più di due mesi, consentendo un cambio di maggioranza che, nelle prospettive in cui ci era stato raccontato, avrebbe dovuto incidere diversamente sulla stesura del Piano. Come sempre, invece, si sta lasciando tutto nelle mani del Governo,

Signor Ministro, non bisogna dimenticare che il *recovery plan* costituisce - sì - una grande opportunità per l'Italia di uscire da una crisi economica scatenata da una pandemia mondiale, ma il - lo sa meglio di noi - sta non già ricevendo concessioni dall'Europa, bensì contraendo un debito di 127 miliardi di euro, che sicuramente lasceremo alle future generazioni e ai nostri figli. Per questo, non possiamo lasciare che sia solo il Governo a decidere cosa si farà su questo Piano. Dobbiamo essere messi nella condizione di sapere quali saranno gli interventi, gli investimenti e le riforme da fare per avere la dotazione finanziaria che il *recovery plan* consente di ricevere.

che riteniamo che sul Piano nazionale di ripresa e resilienza ci siano ancora ampi margini di miglioramento, se però il Parlamento verrà messo nelle condizioni di lavorare.

proposte di risoluzione presentate dal Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia.

in un anno indubbiamente molto difficile, forse il più difficile che il Paese abbia mai affrontato dal dopoguerra a oggi. Stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel, grazie alla scienza e alla ricerca, con la realizzazione, in meno di dodici mesi, di più di un vaccino sicuro ed efficace. Ci troviamo però ancora in una fase molto complessa, in cui è necessario tener duro e abbiamo tutti il dovere di mostrare al Paese unità e responsabilità rispetto a un obiettivo comune, che è quello di uscire dalla crisi sanitaria per tornare alla normalità, perché sulla salute e sulla vita delle persone non possiamo dividerci. Il virus colpisce tutti indistintamente, ma nei momenti di crisi ed emergenza le società affrontano la scarsità di risorse, che amplifica le disuguaglianze e le fragilità e aumenta le distanze tra chi potrà avere un'opportunità e chi non ce la farà. È per questo che dobbiamo ripensare la nostra società alla luce dell'impatto devastante che questa pandemia che questa pandemia ha avuto sulle nostre esistenze, aggravando i problemi strutturali che affliggono il nostro Paese e che per molti anni ci hanno impedito di crescere e allargando il divario tra le persone: un divario di genere, territoriale, generazionale e formativo, un divario di opportunità. L'Italia non può affrontare questo impatto da sola, lo abbiamo sempre detto. Un anno fa il *premier* Draghi pubblicava sul «Financial Times» un manifesto della nuova Europa al tempo del Covid, in cui evocava un cambiamento di mentalità, come durante la guerra. Diceva infatti che dobbiamo sostenerci l'un l'altro come europei, per affrontare questa che è, evidentemente, una causa comune. un richiamo bello, a ritrovare l'autentico spirito dell'integrazione europea, che è fondato sulla consapevolezza che la solidarietà tra Paesi non è un'opzione, ma è l'unica via che abbiamo a disposizione per uscire da questa crisi. Il primo passo di questa strada è stato proprio il Next generation EU, uno strumento da destinare agli Stati per affrontare l'impatto economico e sociale della pandemia, garantendo la crescita, ma anche la capacità di resistere alle crisi future. Per l'ammontare delle risorse, si tratta di un investimento che capita una volta in una generazione e questo significa che tutti noi, qui dentro - so che lo sentiamo tutti nello stesso modo - abbiamo una responsabilità enorme. Credo sia molto giusto dare atto al precedente Governo di aver sottoscritto un'intesa storica, perché, al netto delle risorse, per la prima volta gli Stati hanno deciso di fare debito comune, per finanziare piani contro la recessione e l'Italia è stata il più grande beneficiario di questi stanziamenti. Le uniche condizioni sono la qualità della spesa e le riforme. Dobbiamo rendere però permanente il Next generation EU e cambiare il patto di stabilità, per trasformarlo in un vero patto di sostenibilità sociale e ambientale. Se riusciremo a farlo, avremo messo in sicurezza il Paese per i prossimi anni e avremo rafforzato la logica solidaristica in cui si condividono i rischi e le fragilità, quella logica per cui la protezione sociale dei cittadini e la costruzione di opportunità per ognuno sono centrali, in un'Europa che sia rete di protezione e di possibilità. *(Applausi)*. Crediamo nell'Europa; nell'Europa; da sempre, e non abbiamo mai cambiato idea: lo pensavamo ieri e lo pensiamo ancora oggi; l'Italia senza l'Europa sarebbe più sola e avrebbe meno opportunità e siamo convinti che questo Governo, profondamente europeista, saprà dare il suo contributo a tale progetto. Siamo contenti che chi fino a pochi mesi fa invocava l'Italexit oggi si sia convertito sulla via dell'europeismo, perché non è mai troppo tardi e da questi problemi se ne esce solo se stiamo tutti insieme. Per fare in modo che l'occasione che abbiamo non sia sprecata, questi soldi vanno spesi bene. Spendere bene significa investire sul domani e non su misure per raccogliere consenso oggi; significa giovani, donne, istruzione, formazione, innovazione e lavoro e creare le condizioni che permetteranno al nostro sistema economico di mettere in moto un percorso di crescita, che si traduce in maggiore benessere per i cittadini. Per spendere bene - lo sappiamo - servono le riforme e intrecciare obiettivi con strumenti, e non è un caso che la Commissione europea abbia definito i Piani di ripresa e resilienza come piani di investimento e di riforma. Le riforme sono gli strumenti per garantire l'efficacia e la rapida attuazione degli investimenti, ma anche per superare i nostri limiti strutturali che hanno soffocato la crescita. Velocizzare non significa trascurare trasparenza e legalità e dovremo vigilare e proteggere le tante imprese che stanno sul mercato rispettando le regole. Le riforme servono per fare il bene della società e non per agire contro di essa, per scardinare privilegi e non per mantenere quelli di pochi; pochi; per migliorare la condizione di tutti i cittadini e non solo per favorire quella di alcuni e in particolare - pensiamo che sia tra le priorità serve una riforma della pubblica amministrazione, che non può più essere vista come un ostacolo al cambiamento, ma come un motore per trainarlo. Serve stare al fianco degli enti locali che si troveranno a essere interpreti di tutti questi cambiamenti che sono richiesti e i territori dovranno essere protagonisti. Le riforme non sono semplici atti normativi; sono processi politici, ma anche la chiave di volta per costruire un'Italia più forte e moderna, che sappia stare al passo con gli altri Paesi e che promuova occupazione, crescita sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale. Signor Ministro, per fare le riforme serve essere coraggiosi, lo sappiamo,

i nostri ragazzi vivranno nel mondo della quarta rivoluzione industriale, la più complessa. Dobbiamo metterli nelle condizioni di stare in questo nuovo mondo da protagonisti, di sognare un futuro e di vedere realizzare i loro processi di vita.

L'Italia è anche un Paese che mortifica le donne con tassi di occupazione femminile molto bassi. Senza lavoro non c'è libertà per le donne - ce lo ricorda sempre anche la presidente Valente della Commissione

Sia chiaro: gli investimenti previsti nei Piani di ripresa e resilienza non sono e non possono essere soltanto misure risarcitorie e mirare a ripristinare uno scenario pre pandemia che già ci vedeva tra gli ultimi in Europa. Serve un cambio di passo, a partire da una reale, vera parità salariale, un *welfare* più presente ed efficace, in maniera tale da consentire che le migliori energie della metà della popolazione possano essere liberate. Questa è l'ultima chiamata per modellare finalmente il nostro Paese a misura di due, per definire una nuova grammatica, che non sarà solo negli investimenti, ma nella costruzione di una società più equa, più giusta, perché come ci insegna quello che sta accadendo in alcuni Paesi europei, è dallo spazio pubblico, dalla piena cittadinanza civile e politica delle donne che passa la tenuta di uno Stato di diritto, un Paese quindi più forte e più democratico per tutti. Lo dico con orgoglio: il Senato monitorerà la ricaduta di tutte queste proposte, volendo adottare una vera cultura della valutazione che farà del bene al Paese

un elemento che potrà guidare nelle scelte che, tra qualche giorno, tra qualche settimana, si concretizzeranno nei progetti. Dico subito in premessa

perché credo che il lavoro prezioso - di chi ha votato a favore e di chi magari non voterà a favore, ma comunque ha dato un grande contributo - debba essere la guida attraverso cui concretizzare i progetti. Dico anche un'altra cosa, e ci dobbiamo capire su questo: la Next generation EU è una risposta buona, giusta, finalmente di un'Europa solidale, alla crisi pandemica, ma anche - lo sottolineo,

in un Paese che ha compiuto il salto di qualità e la riconversione ecologica. Per questo non è più tempo di traccheggiare; non è più tempo di passi timidi. È il tempo in cui tutti dobbiamo assumerci fino in fondo,

Non è retorica del cambiamento; sono i fatti. Dobbiamo recuperare rapidamente tutti i problemi, nonché intervenire sui problemi strutturali di questo Paese, come hanno detto moltissimi colleghi; problemi strutturali che certamente ci portavamo da molto tempo, e questo è certamente un problema vero e forte. Diciamocelo chiaramente: parlare genericamente di crescita oggi non significa più nulla. Oggi dobbiamo accelerare perché parte da qui la possibilità del futuro, la riconversione del sistema produttivo, del sistema dei consumi e dei trasporti. Sul punto

in quella direzione e dobbiamo anche sapere che possono esserci dei costi sociali. Tuttavia, siccome abbiamo già tanti problemi occupazionali nelle aree di crisi per fare le riconversioni, bisogna sapere che dobbiamo puntare alla transizione giusta, quindi accompagnare, sapere, incentivare quelli che possono fare di più e disincentivare in altri casi, ma avendo ben chiaro che il fronte sociale dobbiamo sempre tenerlo aperto.

sul Mezzogiorno, su cui tornerò, sulla parità di genere, sulla salute) deve essere verificato, non deve arrecare danni ambientali. Ricordiamoci che l'unità di misura dei nostri progetti è quella.

costruire un piano che non sia un *collage* di microprogetti o magari di sistemi di *bonus* o di incentivi, che servono laddove servono. Dobbiamo avere la capacità di costruire davvero seriamente, con visione del futuro, un impianto strategico che abbia tutte le connessioni giuste, perché le unità di misura sono quelle:

questa legislatura) nella storia per questo, se saremo capaci di impostare un Piano che magari altri continueranno a portare avanti, che abbia questa visione strategica e che abbia la possibilità di cambiare davvero questo Paese.

mi sia consentito un ringraziamento iniziale, come hanno fatto anche altri colleghi, a tutti i parlamentari e a tutti i senatori che nelle Commissioni permanenti, in queste settimane, hanno lavorato per raggiungere oggi questo risultato. un ringraziamento, anche perché non è stato un lavoro facile, ai relatori, presidenti Dario Stefano e Daniele Pesco. Soprattutto, aggiungo un ringraziamento particolare al mio Gruppo parlamentare e a tutti i nostri

pubblica amministrazione, infrastrutture, giovani, donne, lavoro e anche le proposte su Roma Capitale), sono importanti. Quindi, invitiamo il Governo a tenerle in debita considerazione.

assolutamente una cura e quindi è scoppiata la pandemia. L'anno 2020 è stato un anno spartiacque delle nostre vite, delle nostre abitudini e delle consuetudini. Siamo passati da una vita sociale aperta all'isolamento e al distanziamento sociale, in attesa che la scienza, così come ha fatto, con i suoi passi da gigante, trovasse il vaccino, oggi indispensabile per contrastare la malattia. Quanto ci è costato questo anno non vissuto in termini sociali ed economici? Ci è costato tantissimo.

Quindi, il bilancio dell'ultimo anno è apocalittico, una situazione eccezionale che necessita oggi di essere affrontata con strumenti eccezionali. Ecco perché noi oggi siamo Siamo qui ad esaminare le proposte contenute nel più grande Piano di rilancio della storia repubblicana, reso possibile grazie al sostegno e alla condivisione di risorse e obiettivi della nostra casa comune, che si chiama Europa. Next generation EU non può sfuggire al paragone con l'altro grande precedente Piano di rilancio che ha visto il continente europeo protagonista dopo la Seconda guerra mondiale, il Piano Marshall. Quindi, è utile, anche oggi, fare un confronto con il Piano Marshall, perché le analogie non mancano. Entrambi sono progetti di rilancio di rilancio della nostra economia, per far ripartire soprattutto l'economia, nel primo caso, dopo la Seconda guerra mondiale, con il Piano Marshall, e, in questo caso, dopo la pandemia e dopo il coronavirus, con un Piano in grado di mobilitare investimenti ingenti in settori strategici.

di prestiti a fondo perduto che sono bilanciati soltanto da una condizionalità, quella delle riforme strutturali. Il confronto tra i due Piani è sorprendente:

l'opportunità di dare finalmente corpo a tutte quelle riforme che non sono più rinviabili, soprattutto nell'interesse delle prossime generazioni, perché sulle prossime generazioni graverà anche il debito che stiamo contraendo. Per le riforme non possiamo più aspettare ed è necessario, anche con

inefficiente e un controllo puntuale degli sprechi; in tema di commercio, favorire l'accelerazione della transizione digitale, affinché le piccole e medie imprese oggi siano tutte connesse in rete, una rete ultraveloce. Ribadiamo il concetto della spesa da impegnare - oggi il relatore chiedeva anche di più del 34 per cento - per il Mezzogiorno

Per la missione 2 sono importanti una serie di incentivi a fondo perduto, anche di carattere fiscale, per il rinnovo del parco mezzi circolante. Dobbiamo puntare sulla meccanizzazione verde, sull'agricoltura di precisione, sui macchinari di nuova generazione. Da decenni nel nostro Paese manca una politica delle infrastrutture degna di questo nome. È importante connettere oggi tutta l'Italia con l'Alta velocità. *(Applausi)*. È importante oggi migliorare i trasporti regionali, le strade e le autostrade.

e soprattutto nel ridisegnare l'assistenza ospedaliera, potenziando la struttura organizzativa dei reparti in modo da snellire le liste d'attesa. Quindi, occorre intervenire anche sui reparti di aree critiche, sulle sale operatorie e le terapie intensive, stabilizzando nuovi posti letto; soprattutto è necessario l'assistenza domiciliare, creando una rete territoriale per una sanità integrata. Questa è solo una parte di tutte le proposte che sono state oggi accolte nella relazione finale, che - come dicevo - è una sintesi. Però ce ne sono, caro Ministro, tante altre che sono state discusse qui quest'oggi e ieri nella discussione generale in Parlamento. Inviterei il Governo a farsene carico e a valutarle, anche tutte quante insieme.

Sta a noi oggi, classe dirigente in questo momento di questo Paese, sfruttare questa grande possibilità e opportunità: quella di far riprendere l'economia del nostro Paese. Paese. Una classe dirigente che si rispetti oggi non può assolutamente perdere la sua credibilità e, quindi, ha la necessità di puntare dritto allo sviluppo del nostro Paese, alla ripresa dell'economia, alla ripresa della socialità.

Ci tengo ad esprimere, in questa dichiarazione, tutto il senso delle mie parole di ieri. In molti, in questi ultimi tempi, si saranno chiesti come mai la Lega sia entrata a far parte di questo nuovo Governo. La risposta è anche in quello che stiamo facendo oggi.

cosa che abbiamo vissuto sulla nostra pelle da spettatori fuori dal Governo, non potevamo permettere che ancora una volta il Paese fosse penalizzato da questa gestione. Non potevamo e non possiamo permettere, ancora una volta, dopo un anno di pandemia, che questa grande occasione che ci è stata concessa vada sprecata. Ci siamo sentiti in dovere di intervenire: abbiamo voluto, con la nostra dare una forte scossa alle scelte politiche, che erano ormai piatte da mesi. Altrimenti questa triste storia, fatta di sprechi, si sarebbe nuovamente ripetuta. Anche per questo siamo entrati nel Governo; non per il bene della Lega, partito al quale abbiamo dato e daremo sempre il cuore, ma per il futuro dei nostri figli e per l'Italia intera, da Nord a Sud. Certo, sarebbe stato più facile starsene fuori, criticare senza un'alternativa e guardare il Paese affondare. E poi cosa sarebbe restato tra qualche anno? Un Paese commissariato, come la Grecia, dove greca è rimasta forse solo la bandiera. Il *recovery fund* è anche questo: è un impegno, una grande sfida che non si ripeterà mai più, la sfida che tutti hanno chiamato e chiamano il nuovo Piano Marshall. Ciò che noi stiamo facendo oggi è semplicemente ciò che si dice «metterci la faccia» e, visti i tempi che corrono, non è una cosa da tutti. Non solo ci stiamo mettendo la faccia, ma anche il cuore e tanto coraggio. Abbiamo passato le notti discutendo su parole, su frasi, su righe, su passaggi che stravolgevano e sconvolgevano il senso della relazione prodotta dalle Commissioni. Abbiamo ripreso la questione settentrionale, rimarcando la sua grande importanza strategica; abbiamo ripreso la questione, troppo spesso dimenticata, del Centro, senza mai tralasciare l'importanza di un rilancio serio e tangibile che il Sud ancora aspetta da troppi anni. Abbiamo rimesso al centro del discorso le grandi opere: le ferrovie, le strade. Soprattutto abbiamo deciso di portare in Senato e condividere una battaglia storica della Lega: la revisione di quella tartaruga, tutta italiana, che rallenta ogni cosa tocchi, che è il codice degli appalti. Non ci siamo risparmiati nemmeno sull'ambiente, sul *green*, sulla transizione ecologica, sull'elettrico, sull'utilizzo dall'idrogeno verde e dell'idrogeno blu, sulle fonti rinnovabili; lo abbiamo sempre fatto usando criterio e scevri da ideologie. Questa è la Lega, questi siamo noi: il bene dei cittadini sempre davanti ad ogni cosa. Non abbiamo mai fatto mancare il nostro supporto a un lavoro che abbiamo preso in seconda battuta, entrati solo in corsa in questo Piano come nuova forza di maggioranza. Eppure, nonostante le forti tensioni, che più volte i Presidenti che più volte i Presidenti di Commissione - che ringrazio - hanno saputo abilmente placare, oggi abbiamo di fronte una relazione condivisa, per il bene del Paese e degli italiani. mio intervento di ieri ho detto di sentirmi addosso questo impegno come una forma di rispetto per chi ha perso tutto, parenti, amici, lavoro. Oggi mi sento di aggiungere che questo impegno lo dobbiamo agli italiani a casa, che aspettano di ripartire, di riaprire i loro negozi, di riaprire i loro ristoranti, le palestre. Non c'è più tempo da perdere, non c'è più tempo da sprecare in giochi di palazzo. *(Applausi)*. Il nostro dovere Il nostro dovere è dare risposte e mettere al centro dell'agenda politica solo il bene della nostra gente. Questa triste pandemia sembra non finire più; ogni giorno ci troviamo a lottare contro di essa e a cercare di dare delle risposte. Il problema è che alle volte è difficile anche dare delle risposte. Il nostro dovere è spendere tutte le energie rimaste, dopo più di un anno, per far sì che il Paese riparta con slancio e determinazione, non appena potremo riaprire tutto. Per tutti questi motivi, la Lega esprimerà un voto favorevole sulla proposta di risoluzione della maggioranza, con la certezza che il Governo terrà conto delle linee guida condivise da tutti.

Credo di interpretare il sentimento di tutta l'Assemblea nel far giungere al senatore Candiani

Signor Presidente, ministro Franco, Governo, colleghi, abbiamo vissuto per anni come se avessimo infinite risorse a disposizione. Abbiamo vissuto pensando esclusivamente al presente, senza ricordare il passato e senza volere o sapere immaginare il futuro. E in questo presente il nostro unico obiettivo era la produzione, una produzione che doveva crescere di anno in anno. cento di ciò che produciamo, però, diventa rifiuto e così abbiamo messo a rischio interi ecosistemi, la sopravvivenza di specie animali e vegetali; abbiamo favorito il diffondersi di malattie come le zoonosi, di cui fa parte la Covid, e quindi anche l'incubo che viviamo da un anno a questa parte è una conseguenza del nostro modo di vivere. Il nostro pianeta, il nostro buon pianeta, è in pericolo; non c'è più tempo da perdere. Un rimedio lo abbiamo: la chiave di volta deve essere la transizione ecologica che non va vista come una ciliegina da aggiungere alla torta, alla fine e se c'è tempo. Per mettere in atto la transizione ecologica abbiamo uno strumento straordinario: gli oltre 200 miliardi di euro affidati all'Italia grazie all'immenso lavoro del presidente Giuseppe Conte. Grazie a questi fondi la transizione ecologica può diventare la torta. Però dobbiamo avere il coraggio di intraprendere riforme che siano vere e proprie prove per costruire l'Italia del 2050, a partire dall'ambiente, che è la nostra prima stella e che deve essere la stella di tutti. risoluzione che abbiamo redatto abbiamo chiesto di incrementare i fondi in ricerca e sviluppo destinati all'economia circolare, di aumentare i progetti di forestazione urbana, di prevedere percorsi universitari e post-universitari in transizione ecologica. Vogliamo poi rafforzare il binario salute e ambiente che per noi è fondamentale: non c'è salute in un mondo malato. Per rafforzare questo binario dobbiamo innanzitutto lavorare sulla connessione dei dati tra il sistema sanitario e quello di raccolta dei dati ambientali; solo così potremo mettere in atto la prevenzione, che è ancora l'arma più potente che abbiamo per sconfiggere le malattie, malattie, intesa non solo come prevenzione primaria (corretti stili di vita), ma soprattutto come prevenzione secondaria (diagnosi precoce). In Italia l'adesione agli *screening* oncologici è ancora troppo bassa e va rafforzata, così come vanno potenziati gli investimenti per garantire che ci siano *screening* neonatali per patologie genetiche e metaboliche, a partire da quella legge importantissima voluta dalla nostra vice presidente Taverna. Al centro della sanità che immaginiamo, di questa rivoluzione dei servizi alle persone, noi mettiamo però il territorio, la medicina territoriale, che è stato l'anello debole anche nella gestione della pandemia. Rafforzare il territorio vuol dire utilizzare gli strumenti di telemedicina, costruire le case e gli ospedali di comunità che devono fare da filtro ai grandi nosocomi. Fino ad oggi abbiamo concentrato le cure tutte in ambito ospedaliero, anche per i malati cronici e oncologici. Ricordo ancora con estrema tristezza il racconto di una delle mie più care amiche che ogni venti giorni doveva recarsi a fare la chemioterapia all'ospedale di Pozzuoli che distava 20 chilometri. Mi raccontava di come i viaggi di ritorno dopo la terapia potessero durare anche ore perché doveva fermarsi di continuo per i conati di vomito indotti dalla terapia. Rafforzare il territorio vuol dire non sottoporre più i pazienti allo stress del viaggio, del dover abbandonare abbandonare la propria casa, vuol dire mettere al centro la persona. In questa pandemia abbiamo anche toccato con mano come non sia garantito su tutto il territorio nazionale lo stesso diritto di accesso alle cure. Ecco perché chiediamo di rivedere il Titolo V, dando più potere di indirizzo allo Stato centrale. Le Regioni devono essere gli enti attuatori, ma non devono poter derogare a quelle che sono le disposizioni che provengono dal Governo. differenze territoriali in tanti ambiti, dalle infrastrutture, ai trasporti, ai servizi alla persona; ecco perché una fetta importante dei fondi è indirizzata proprio alla coesione territoriale. L'Italia non può ripartire se non riparte il Mezzogiorno. Il Mezzogiorno deve ripartire dalla valorizzazione delle risorse umane. Oggi i giovani del Sud devono emigrare per necessità e non per scelta. Faccio solo l'esempio dei dottorati; per formare un dottorato l'Italia spende 400.000 euro, ma solo uno su tre dei dottorati che formiamo può restare nel nostro Paese, soprattutto se proviene dalle Regioni del Sud. Questo vuol dire che noi stiamo regalando i nostri investimenti agli altri Stati, stiamo facendo degli investimenti a perdere. Valorizzare il capitale umano vuol dire permettere alle donne, soprattutto del Sud, di poter meglio conciliare la vita familiare e la vita lavorativa; ecco perché chiediamo di estendere il tempo pieno alle scuole primarie e secondarie su tutto il territorio nazionale di costruire più asili nido. In Europa il 33 per cento dei bambini frequenta un asilo nido. In Italia solo il Nord-Est raggiunge questo valore, mentre il Sud e le isole sono fermi al 12 per cento. È un aspetto 40 miliardi dei fondi stanziati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sono indirizzati alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica che non vuol dire solo utilizzare tecnologie più innovative, ma anche riorganizzare i processi per offrire migliori servizi ai cittadini. Presentiamo poi la nostra nuova visione di impresa con misure straordinarie e rivoluzionarie come l'ecobonus 110 per

a tanti nostri cittadini di poter ristrutturare la propria casa, di trasformarla in modo ecosostenibile. Mi soffermo infine sull'istruzione e la ricerca, due temi che ci stanno molto a cuore. La scuola e lo studio devono un diritto di tutti e non un privilegio di pochi. rafforzando il diritto allo studio innalzando la soglia ISEE al di sotto della quale non si pagano le tasse universitarie da 13.000 a 23.500 euro. Questo vuol dire che permetteremo a tutti gli studenti meritevoli che provengono da famiglie non particolarmente avvantaggiate di poter intraprendere percorsi di studi universitari, di realizzare il proprio sogno, di mettere a frutto il proprio talento. Infine, la ricerca. Oggi l'Italia è al ventisettesimo posto nell'area OCSE per investimenti in ricerca e sviluppo, con solo l'1,4 per cento del PIL dedicato a questi settori, di cui appena lo 0,5 per cento proviene da investimenti pubblici. siamo all'ottavo posto in termini di produttività. Questo vuol dire che abbiamo delle eccellenze che non sappiamo valorizzare. Signor ministro Franco, nell'annunciare il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle alla proposta di risoluzione di maggioranza, voglio ribadire che noi oggi gettiamo le fondamenta del futuro, di un'Italia del futuro che sia più competitiva, che conquisti il centro del palcoscenico europeo. È necessario partire dalla transizione ecologica per costruire l'Italia del 2050. Diceva San Francesco di partire da ciò che è necessario, fare ciò che è possibile per poi ritrovarsi a realizzare l'impossibile. *(Applausi)*.

c'è la misura della vostra poca democrazia, ma noi di L'alternativa c'è in questi tre minuti sapremo dirvi che cosa state facendo e che cosa avremmo dovuto fare nell'interesse del Paese. Quanto a ciò che state facendo, voi oggi approvate una relazione fumosissime pagine che non dicono affatto al Governo come spendere i soldi del Piano, e di fatto consegnate una delega in bianco al Governo delle banche, delle *élite* e degli interessi sovranazionali. Che cosa invece avremmo dovuto fare nell'interesse del Paese? A fronte della scarsità delle risorse, il Parlamento avrebbe dovuto assumersi la responsabilità e il coraggio delle scelte; avrebbe dovuto graduare le priorità del Governo e dire di no alle grandi opere inutili, alle cattedrali nel deserto come il ponte sullo Stretto di Messina; sì alla messa in sicurezza, all'efficientamento energetico e all'ottimizzazione delle infrastrutture esistenti; sì al potenziamento della scuola pubblica e della sanità pubblica e non di quelle private; sì agli aiuti ai piccoli imprenditori, ai commercianti e agli artigiani; no ai regali ai grandi gruppi societari; sì alle assunzioni dei giovani nella pubblica amministrazione; no alle consulenze milionarie a società esterne; sì all'ingresso dello Stato in settori strategici dell'economia come l'acciaio o la farmaceutica e alla realizzazione di una banca pubblica per gli investimenti. Ma di tutto questo nella vostra vacua e verbosa relazione non c'è traccia, e il poco che c'è è annacquato tra centinaia di petizioni di principio che sono state inserite alla rinfusa e contrastano le une con le altre. Per questi motivi L'alternativa c'è, sul cui riconoscimento come componente lei, presidente Casellati - che sta parlando e non mi ascolta -, e voi, membri della Giunta per il Regolamento, siete dolosamente inadempienti,

un segnale come un faro nella notte, e accerterà che in questo simulacro di Parlamento, di fronte alla marea montante dell'omologazione, un nucleo di opposizione e di resistenza c'è.

Signor Presidente, onorevoli senatori, signori del Governo, sono due gli aspetti emersi dal confronto tra i sindaci aderenti alla rete *recovery* Sud su cui voglio porre l'accento e che mi portano ad annunciare anche a nome loro la mia astensione. Il primo riguarda le risposte da dare nell'immediato ai cittadini. È chiaro che i fondi del *recovery*, pur rappresentando una potenziale svolta, non hanno risvolti immediati. Per questo chiediamo un'azione concreta che possa dare respiro e fiducia ai tanti cittadini che da troppo tempo sono fermi a causa della crisi. Il secondo aspetto è che le linee di cui stiamo discutendo sono ancora troppo generiche. Come già sancito dalla Camera dei deputati, nella relazione della V Commissione, il *recovery* deve essere destinato e utilizzato al fine di realizzare la coesione sociale, economica e territoriale del nostro Paese, anche in ossequio all'articolo 117 della Costituzione. La rete *recovery* Sud ha chiesto, per questo motivo, di redistribuire i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza secondo i criteri in base ai quali sono stati stanziati dall'Europa: popolazione, PIL *pro capite*, tasso di disoccupazione. Secondo questi parametri, al Sud dovrebbe andare almeno il 60 per cento delle risorse del *recovery plan.* Apprezziamo l'attenzione del ministro Carfagna, che ha ricevuto e ascoltato una nostra delegazione. Ringraziamo il sottosegretario Nesci che ci ha ascoltato e siamo felici di aver avuto la disponibilità di un incontro anche da parte del ministro Bonetti. I sindaci della rete *recovery* Sud, però, per avere fiducia nel Governo, attendono misure concrete e sono pronti a mobilitarsi per chiedere che sia dato al Sud ciò che spetta al Sud. In attesa di valutare nel merito i provvedimenti che saranno assunti dall'Esecutivo, ribadisco la mia volontà di astenermi.

una importantissima parte relativa alla biodiversità e al mare. E questo è anche e soprattutto grazie a me, che mi sto battendo da anni. anni. Le associazioni ambientaliste e il mondo della ricerca scientifica stanno parlando al Governo e chiedono che gli impegni del Parlamento vengano soddisfatti e quindi che il Governo possa utilizzare il primo pilastro, quello della transizione verde, compresa la biodiversità, come la parte più importante, visto che l'Italia è l*'hotspot* della biodiversità nel mondo.

Per questo motivo, attendo che il Governo faccia la sua parte e inserisca il tema del mare: se si parla di cambiamenti climatici, si deve parlare di mare e di economia blu.

il Parlamento chiede al Governo di assumere non ci arriveremo mai, perché è stato estremamente prudente

Non si è detto che serve una moratoria con il *capacity market*. Non si è detto assolutamente che l'idrogeno blu è stato bocciato dall'Europa e si sono chiesti degli investimenti in quel settore

mai, sveliamo il vostro inganno. I soldi di Bruxelles hanno un duplice inganno: il primo dei quali dato dalle stringenti condizionalità europee, visto che dovremo seguire una *road map* precisa. Il secondo inganno è che tutti i denari che ci arrivano andranno restituiti, anche quelli cosiddetti a fondo perduto. Insomma, di materno l'Europa non ha proprio nulla, nonostante al *recovery* sia attribuita una funzione catartica e consolatrice, uno *shampoo*. Il PNRR è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco, una mamma enorme, una mamma in bianco. E allora sciacquo, sciacquo; una sciacquata *green* e ambientalista, in nome della eco-sostenibilità tesa a uno spostamento verso l'elettrico e l'idrogeno. Dite che ad Alitalia arriveranno tanti soldi da spendere. Certo, soldi da spendere a debito per favorire le economie degli altri: tedeschi e cinesi in testa perché saranno loro a venderci l'elettrico. Riassunto: a noi i debiti dei prestiti, agli altri i profitti. Ma lo *shampoo* ecologista deve andare avanti ed essere spinto. C'è chi crede che sia meglio quello senza canfora, anche se i migliori sono i più cari perché sono antiforfora. La schiuma è una cosa sacra che pulisce la persona meschina, abbattuta e oppressa. Infatti, ripulita, la mandiamo sui monopattini, che sono l'oggetto che più impatta sulle emissioni di CO2; dalla produzione allo smaltimento. Stiamo comprando oggetti cinesi, dannosissimi per l'ambiente, dalla vita brevissima, in nome dello *shampoo* ecologista. Che dire dei porti *green*? L'Europa, con una lettera della solita Vestager, vuole privatizzare i porti italiani, ma non vede il *dumping* anche ambientale dell'Olanda. Forse non sapete quanto inquinano le migliaia di navi cargo che arrivano a Rotterdam, anche pieni di merce contraffatta dalla Cina. Ma «sciacquo, sciacquo!». A proposito, in tutto questo sciacquo, avanza qualcosa per abbassare le bollette? Se infatti consumo energia pulita, allora perché devo pagare gli oneri di sistema? Abbiamo le bollette tra le più care d'Europa, ma che importa? «Sciacquo, sciacquo e poi... *phon*!». Aveva ragione Gaber: «con tutte le libertà che avete, volete anche avere la libertà di pensare?». Meglio di no, altrimenti poi scoprireste la verità.

Signor Presidente, i tempi della politica non coincidono con le esigenze delle piccole e medie imprese, delle attività commerciali, di bar, alberghi e ristoranti e con le condizioni peggiorate dalla tragedia pandemica per le famiglie. Abbiamo avuto oltre 800.000 disoccupati in più. Secondo l'osservatorio sui bilanci dei commercialisti, su 830.000 società, che fatturano 2.700 miliardi di euro,

Tra marzo 2020 e gennaio 2021, a fronte di finanziamenti alle imprese, assistiti da garanzie pubbliche per circa 140 miliardi di euro, il flusso dei prestiti alle imprese è stato di oltre 420 miliardi

che rappresentano l'ossatura di un Paese che è la seconda manifattura europea, rischia di non riaprire i battenti, con l'aggravante della ricetta neoliberista uscita dal G30, secondo la quale per battere la pandemia occorre applicare il darwinismo in economia, lasciando al loro destino le imprese *zombie*, soprattutto le piccole, contribuendo così alla desertificazione delle città. In questa situazione disastrosa per i conti pubblici, a Pasqua si impediscono gli spostamenti tra le Regioni italiane, offrendo la possibilità di andare in vacanza all'estero, offrendo una ghiotta occasione di incrementare il turismo ai nostri diretti concorrenti, mentre i nostri stabilimenti balneari gli albergatori chiudono i battenti. Per offrire la possibilità di sopravvivenza a molte attività economiche, alberghiere e del turismo occorre una moratoria di quindici o vent'anni sui prestiti contratti con le banche, che non potranno essere onorati con le chiusure forzate, essendo irrisori i contributi sulle perdite annuali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

domani, 2 aprile, si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, che rappresenta un momento di meditazione e riflessione molto rilevante. La legislazione più recente sui disturbi dello spettro autistico ha fatto registrare notevoli passi avanti, insieme a un'opinione pubblica sempre più consapevole delle insidie e delle complessità connesse a questa tipologia di disturbi. L'approvazione della legge n. 134 del 2015, l'istituzione dei fondi statali appositamente dedicati e l'inserimento nei LEA dell'erogazione pubblica delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento, con l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, costituiscono certamente un buon punto di approdo. Tuttavia, a partire da oltre un anno, il contesto pandemico ha rivoluzionato la quotidianità di chi soffre di disturbi dello spettro autistico, aggravando spesso situazioni basate su un equilibrio assai precario. L'emergenza da Covid ha inciso profondamente sullo *status* di ogni essere umano, ma ha intaccato ancora più in profondità la coscienza delle persone più fragili e delle loro famiglie. Il *lockdown* del 2020 e le misure di contenimento prese per contrastare il Covid non hanno permesso ai ragazzi con disturbi dello spettro autistico di poter trovare quei momenti di socialità e svago che sono per tutti indispensabili. Abbiamo dunque il dovere morale e sociale di aiutare ancora di più chi ha attraversato enormi difficoltà in un momento storico che ha messo in ginocchio l'intero Paese. In questo momento in cui si intravede una luce in fondo al tunnel voglio anche mandare un messaggio di speranza, perché molte iniziative della società civile promuovono l'inclusione, soprattutto in tempi così avversi. Nella Provincia di Salerno si stanno sviluppando numerosi progetti basati sulla comunicazione aumentativa e alternativa, con l'obiettivo di aiutare chi ha difficoltà a utilizzare i più comuni canali comunicativi orali e scritti. Un'associazione in particolare, «Insieme si può Sarno», sta promuovendo l'utilizzo del menù CAA, uno strumento di inclusione sociale grazie al quale il menù di un ristorante o di una gelateria diviene accessibile anche a un ragazzo o a una ragazza che soffre di disturbi dello spettro autistico. È un'iniziativa veramente lodevole in questo momento storico in cui chi è affetto da disturbi autistici può accusare maggiormente lo stress dovuto all'applicazione delle misure contro la pandemia. Con la legge di bilancio per il 2021 sono aumentate di 50 milioni di euro le risorse del fondo per l'autismo, definendo anche la ripartizione percentuale per i singoli interventi. Fermo restando quanto di buono è stato fatto finora, credo sia quanto mai opportuno aumentare ulteriormente le risorse del fondo. Già a partire dall'esame... *(Il

istituita per richiamare l'attenzione sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e sulle difficili problematiche delle loro famiglie, cioè di chi vive e convive ogni giorno con quella realtà, con quella realtà, voglio riportare l'esempio di chi cerca di affrontare con impegno quotidiano e con profondo spirito di solidarietà tutti i profondi risvolti, anche sociali, di questa disabilità. Ad Arzano, un Comune napoletano, è nata una realtà per minori e adulti autistici, una vera e propria oasi di solidarietà e di condivisione per persone nelle quali - come ben sappiamo - l'aspetto preponderante della loro disabilità è rappresentato dalla chiusura verso il mondo esterno. La struttura è nata grazie alla caparbietà e al coraggio di Antonio, padre di un bambino con spettro autistico, che ha abbandonato la sua attività imprenditoriale, convertendo la propria struttura lavorativa in un centro polifunzionale per ragazzi disabili, dove ospita l'associazione "Noi possiamo" ONLUS. Nel centro, bambini e ragazzi imparano a svolgere diverse attività manuali, come fare la pizza, o giochi e attività sportive con impegni multipli, al fine di coinvolgerli in maniera completa, stimolare la loro partecipazione, provare a rompere quel muro grigio che li isola e sembra separarli e allontanarli dagli altri. È il tentativo sofferto e partecipato di chi è in prima linea, di chi vive in prima persona tutte le difficoltà e le complesse problematiche della gestione di quei bambini e tocca con mano ogni giorno le conseguenze negative della cattiva organizzazione - ancor più in questi momenti di emergenza sanitaria pandemica delle strutture che dovrebbero prendere in carico soggetti che difficilmente riescono a comunicare o a relazionarsi verbalmente, ma lo fanno con suoni e gesti.

fare qualcosa per il proprio figlio e anche per i tanti ragazzi come lui, creando per loro una vera e propria opportunità, lo sport e il gioco come mezzo di integrazione sociale; stimolare tutte le attività sensoriali, coinvolgendole in un percorso riabilitativo in cui lo spirito di solidarietà e il sostegno delle famiglie spesso lasciate sole offrono opportunità dal profondo significato umano e sociale. L'autismo non è contagioso, l'ignoranza sì. Signor peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio e usurpazione di funzioni pubbliche sono alcuni dei reati commessi più frequentemente nel nostro Paese che causano gravi malfunzionamenti degli apparati amministrativi. I costi economici della corruzione sono considerevoli, tanto da determinare una grave perdita di competitività del Paese e pericolose conseguenze sul bilancio dello Stato. Dal gennaio 2021 gli indagati per corruzione sono 164, ossia 2,5 al giorno, mentre gli accusati di mafia, che spesso intreccia i suoi affari con gli apparati degli enti pubblici, sono ben 503, quasi otto al giorno, con un patrimonio di beni confiscati alle mafie pari a 973 milioni di euro in totale dall'inizio dell'anno. L'ultimo *report* pubblicato da Libera sullo stato dell'attuazione della legge sui beni confiscati alle mafie purtroppo rivela che, su 1.076 Comuni monitorati destinatari di beni immobili sequestrati, ben 670, pari al 62 per cento del totale, non pubblicano l'elenco sul loro sito Internet, così come previsto dalla legge. Il primato negativo spetta al Sud, con 392 Comuni inadempienti; segue il Nord Italia con 213 Comuni e il Centro con 65.

Tenuto conto che la pubblicazione di detti elenchi sarebbe obbligatoria per legge e consentirebbe ai cittadini di inoltrare richiesta per il riutilizzo a scopo sociale di una tale mole di patrimonio; considerato inoltre che l'inadempienza da parte delle amministrazioni locali responsabili dei beni confiscati a loro assegnati ha il sapore dell'omissione, quando non della connivenza, chiederemo al Ministro quali azioni intende mettere in atto al fine di rafforzare e rendere efficaci i controlli sulla trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione. Presidente, intervengo per dire anche a quest'Aula che gli insediamenti industriali della Basilicata non si toccano, ma si tutelano. Faccio due esempi attuali e veloci. Tfa (ex Firema) di Tito: 35 dipendenti, commesse in abbondanza nella manutenzione delle motrici e dei treni. Eppure, la proprietà vorrebbe traslocare maestranze e produzione in quel di Caserta. È un'ipotesi che per noi non esiste, assolutamente. Pretendiamo che si porti il numero dei dipendenti a 70-80, per dare stabilità a questa importantissima fabbrica. L'altro esempio è Stellantis di Melfi, già FCA, già Fiat: 7.172 dipendenti diretti, 4.505 dell'indotto. Apprendiamo, in questi giorni tristi e difficili, che, dal 2 al 12 aprile, ci sarà la cassa integrazione. che sono state tagliate drasticamente spese per servizi, mensa, riscaldamento, pulizie tecniche e civili e che già questo taglio ha comportato diversi licenziamenti. Apprendiamo che sarebbe volontà dell'azienda di chiudere una linea, aperta soltanto due anni fa, dove si è prodotta la Jeep Compass. Noi apprendiamo, ma vorremmo che parlasse l'azienda, che sta tacendo e non sta rispettando i lavoratori. Dica, quindi, ai lavoratori quali sono le sue intenzioni, ma soprattutto faccia in modo di mantenere tutti gli impegni che ha assunto alcuni anni fa. La Stellantis di Melfi è stata e deve rimanere punta di diamante nell'*automotive*. Sono certo che Regione e Governo faranno la loro parte. L'azienda e la proprietà facciano altrettanto per garantire stabilità alla fabbrica, serenità ai lavoratori e prospettiva a quell'importante territorio. Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, intervengo sul recente decreto del direttore generale della pubblica sicurezza e capo della polizia, che ha disposto la soppressione del posto di polizia ferroviaria di Campobasso. soppressione rappresenta l'ennesimo atto di depauperamento di un territorio che, negli ultimi anni, ha già pagato dazio, fin troppo abbondantemente, in termini di tagli di servizi e presidi, da parte di tutti i Governi che si sono succeduti alla guida del Paese. Tale provvedimento - come evidenziato nei mesi scorsi, anche dalle parti sindacali - discende da una cronica mancanza di personale di polizia, alla quale bisognerebbe rispondere con un apporto di nuove leve, ancora maggiore rispetto a quanto si sta oggi garantendo, non certo con una soppressione di uffici di polizia, con relativo pregiudizio della sicurezza dei cittadini. L'ufficio Polfer, di cui è prevista la chiusura, ha competenza su quasi tutta la rete ferroviaria della regione Molise, Provincia di Isernia compresa. Proprio la precedente chiusura del posto Polfer di Isernia ha favorito la nascita della microcriminalità, con episodi di furto, asportazione di rame, delinquenza, spaccio, prostituzione, violenza e degrado. stiamo parlando di Isernia, una delle città più tranquille d'Italia, che ha visto cambiare il tenore della vita dei propri abitanti. Evidentemente, non si è voluto fare tesoro di quanto accaduto nella provincia pentra e si è deciso di condannare anche i campobassani al degrado del proprio centro cittadino. L'invito, quindi, è di rivedere subito questa decisione, la quale, peraltro, non comporta alcun risparmio economico per le casse dello Stato. Infatti, i locali dove ha sede il posto di polizia ferroviaria di Campobasso sono di proprietà delle Ferrovie dello Stato, come anche ciò che ruota all'interno della struttura in uso alla polizia ferroviaria. Economicamente, quindi, il taglio è pari a zero. La soppressione del presidio ferroviario è l'ennesima spoliazione ai danni di un territorio periferico che evidentemente viene considerato, erroneamente, meno a rischio di altri. Non possiamo, però, permetterci di mettere a repentaglio la sicurezza dei viaggiatori e delle reti ferroviarie in generale. Quindi, chiedo con forza al Governo, al Ministro dell'interno e al nuovo Capo della polizia, di ritornare sulla decisione. Il Molise e i molisani meritano rispetto e, finché la Regione Molise esiste, lo Stato non può e non deve abbandonarla.